Chiarissima Presidente, ho l'onore di comunicarle, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 87 del 1953,

Nella seduta di oggi sarà discusso il decreto-legge proroga emergenza Covid-19, già approvato dalla Camera dei deputati, in ordine al quale il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia. La settimana dal 28 settembre al 2 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge sul sostegno e il rilancio dell'economia e alle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il calendario dei lavori dal 5 all'8 ottobre prevede lunedì 5, a partire dalle ore 12, la discussione del decreto-legge sul sostegno e il rilancio dell'economia e nei giorni successivi il Rendiconto dello Stato 2019 e l'assestamento 2020, nonché la discussione generale della legge di delegazione europea 2019 e delle connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. 8 ottobre avrà luogo la discussione sulla relazione delle Commissioni riunite 5a e 14a sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alle ore 18,30 di oggi è convocata la Giunta per il Regolamento per avviare l'*iter* di modifica del Regolamento del Senato, a seguito dell'esito del *referendum* costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

deliberata il 31 gennaio 2020. Il provvedimento comprende inoltre disposizioni sul rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza. Il decreto-legge, dopo l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, si compone di quattro articoli e un allegato. A causa dell'estensione fino al 15 ottobre dello stato di emergenza, autorizzata dalle Camere con risoluzioni del 28 e 29 luglio 2020 e deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, è sorta l'esigenza di prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 marzo 2020, che hanno disciplinato rispettivamente l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica. l'articolo 1, comma 1, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, misure tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, allo scopo di contrastare i rischi sanitari da Covid-19. inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il comma 1-*bis,* inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica la lettera *l)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, con l'obiettivo di escludere dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche medico-scientifiche e di educazione continua in medicina. Il comma 2, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, estende al 15 ottobre 2020 l'applicabilità delle misure previste da quel provvedimento. Ricordo che quel decreto-legge (cosiddetto decreto riaperture), pure in continuità con gli strumenti predisposti dal decreto-legge n. ha segnato l'avvio di una nuova fase, contribuendo a delineare una nuova cornice normativa dove le misure differenziali si rivolgono prioritariamente a specifiche aree del territorio sulla base dell'evolversi dei dati epidemiologici. Il comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre

e al 14 settembre 2020), prevedendo che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Si tratta prevalentemente di misure attinenti alla materia sanitaria, oltre che a quelle del lavoro, della scuola e dell'università, contenute in provvedimenti d'urgenza adottati in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra le misure prorogate, ricordo in particolare quelle concernenti l'assunzione degli specializzandi; il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie

con disabilità e per i lavoratori immunodepressi; la continuità della *governance* degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dell'emergenza; la continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale; le attribuzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto all'emergenza sanitaria; la sperimentazione e l'uso compassionevole dei farmaci con riferimento a pazienti affetti da Covid-19; l'accelerazione dell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica. Durante l'esame alla Camera dei deputati è stato aggiunto all'allegato il n. 30-*bis,* ai sensi del quale sono prorogati dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure previste all'articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, 34 (cosiddetto decreto rilancio), relativo alla proroga di ulteriori novanta giorni dei piani terapeutici in scadenza nel periodo dell'emergenza epidemiologica in corso. I piani terapeutici interessati si riferiscono a specifiche patologie che includono ausili e dispositivi monouso e protesici. La proroga si rende necessaria al fine di ridurre il rischio di infezioni da Covid, limitando l'affluenza negli ambulatori specialistici per ottenere il rinnovo dei piani in questione. Ai sensi del comma 4, viene poi precisato che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato, sebbene connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. Il comma 5 dispone che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. da adottarsi sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una Regione o alcune Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020. A tale proposito, si ricorda che il 7 agosto scorso è stato emanato un nuovo decreto del Presidente per il contenimento del contagio, con efficacia fino al 7 settembre, e che il 7 settembre è stato emanato un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia valido fino al 7 ottobre prossimo. Il comma 6 stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Ricordo che attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta; viene la durata massima, che rimane pertanto di quattro anni per il primo incarico più un massimo complessivo di ulteriori quattro anni, prevedendo al contempo la possibilità che vi siano più provvedimenti successivi di rinnovo dell'incarico anziché uno solo. Nella relazione illustrativa del decreto si evidenzia che la disposizione introduce un elemento di flessibilità per garantire le diverse situazioni e i possibili contesti, come ad esempio l'attuale stato di emergenza sanitaria, la continuità e la funzionalità della guida degli apparati di *intelligence.* possibili pregiudizi in un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale. Aggiungo una qualità di questo tipo di norma: in tutte le funzioni dello Stato che debbano presentare una garanzia di terzietà penso per esempio alla Presidenza della Repubblica o alle *Authority* di controllo - la durata prevista per i loro mandati è sempre più lunga di quella della legislatura, questo a garanzia dell'indipendenza di queste cariche, esattamente come noi richiediamo a coloro che difendono la nostra sicurezza un'indipendenza dalla possibile influenza delle maggioranze delle quali Proprio per dare conto di queste disposizioni, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il titolo del decreto-legge in esame è stato integrato. L'articolo 1-*bis* inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati introduce una disposizione di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020 si applichino nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge n. 33 del 2020. Deve essere infatti verificato il coordinamento di alcune misure di contenimento all'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con le misure previste dal decreto legge n. 33, di ambito e portata più circoscritti, posto che il provvedimento proroga al 15 ottobre l'applicabilità degli interventi previsti da entrambi i decreti.

comma 16 del decreto-legge n. 33 consente alle Regioni di introdurre misure sullo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle statali. L'articolo 2, modificato dalla Camera, prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento. Nel corso dell'esame in Commissione, non sono state apportate modifiche. È stato tuttavia approvato all'unanimità un giusto ordine del giorno a favore dei lavoratori fragili: l'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 prevedeva infatti fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti disabili gravi, nonché per i lavoratori in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Poiché tale disposizione non è stata prorogata dal decreto-legge in esame, per la necessità di individuare le idonee coperture finanziarie, con l'atto di indirizzo in questione si impegna il Governo a prorogarla, anche in via retroattiva, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica. Infine, Presidente, una sola considerazione più politica su questo decreto, che è stato seguito lungo queste settimane da vivaci discussioni, se non da polemiche, sull'opportunità di proroga dello stato emergenza. Anche in occasione della discussione generale qui in Senato si è discusso se vi fossero o no i presupposti di fatto per dichiararne proroga. Credo che l'evoluzione dei dati epidemiologici e il quadro mondiale della pandemia, con intere Nazioni, quando non continenti interi, alle prese ancora con numeri di contagio tanto elevati, renda evidente oggi l'opportunità di prorogare modalità che consentano una rapida ed efficace risposta, sposando l'ottica ovviamente della massima flessibilità al mutare delle condizioni epidemiologiche, che non è solo la *ratio* di questo provvedimento, ma che in questi mesi si è dimostrata strumento efficace nella difficilissima sfida contro il Covid-19.

un provvedimento che ha per presupposto la sussistenza dello stato di emergenza. Da parte mia è forte una sensazione di *déjà vu,* mi sembra di tornare indietro di alcuni mesi; tuttavia, lo stato di emergenza - lo sappiamo tutti - ormai non è più sussistente. Attenzione, prima che qualcuno possa obiettare che io mi stia iscrivendo al *club* dei negazionisti, dico che io guardo i numeri che vengono riportati dai giornali: il «Corriere della Sera», che in questi mesi si sta dimostrando un buon sostenitore di questa maggioranza, ha scritto con grande onestà intellettuale per questa parte

Ciò significa che se oggi un alieno ignaro della nostra storia scendesse sulla terra (consentitemi una battuta, durante questa legislatura è successo di tutto e credo che manchi solo lo sbarco degli alieni)

si continua a insistere su questo tema, quando fior di costituzionalisti hanno chiarito che non vi è necessità di mantenere in essere questo stato, anche perché l'eventuale recrudescenza - Dio non voglia - della pandemia potrebbe in poche ore essere fronteggiata con una nuova dichiarazione di stato di emergenza. Quello che mi preoccupa è che noi verremo chiamati ancora una volta a votare la fiducia, a lavorare per la conversione di un decreto-legge quando questo Paese avrebbe bisogno di altro, ad esempio di mettere al lavoro con urgenza delle Commissioni, possibilmente delle Commissioni speciali aperte - quelle sì

di ammettere il fallimento di quest'azione politica e tornare ai propri lavori con dignità, piuttosto che continuare su questa strada. Ebbene, mi chiedo

ma quei soldi si comporteranno come della benzina versata in un serbatoio bucato, perché senza riforme urgenti non saremo in grado di spendere in modo efficace quelle risorse, non saremo in grado di consentire al Paese di ripartire. In questo momento è allo studio, come sappiamo, la riforma del processo civile e del processo penale. Abbiamo un Presidente del Consiglio che è un sostanzialista: insegna, come me, diritto civile. Ora, posso capire che un processualcivilista - è comprensibile - veda nella riforma del processo la panacea di tutti i mali; ma chi conosce il diritto sostanziale sa che il rito è al servizio della sostanza, e se le norme sottoposte all'*iter* processuale sono confuse, caotiche e contraddittorie, non c'è riforma che possa migliorare la situazione. Ma non c'è solo il problema della giustizia civile e di quella penale; c'è anche il problema della giustizia amministrativa, perché i giudici amministrativi sono alle prese (e i cittadini con loro) con un ordinamento amministrativo caotico. Quando servono oltre 70 autorizzazioni - vado a memoria, quindi sicuramente sbaglierò per difetto - per avviare un'attività commerciale, non c'è finanziamento, non c'è *recovery fund* che possa incentivare il giovane (e sono i giovani le nostre risorse) ad avviare un'attività d'impresa. Fate molta attenzione: state barattando la vostra sopravvivenza in questo Parlamento con il futuro del nostro Paese. *(Applausi).* Abbiate il coraggio di guardare in faccia la realtà. Quest'Assemblea è composta da persone di grandi competenze; l'errore sta nel credere che il *vulnus* del Paese risieda nel funzionamento del Parlamento. Il Parlamento ha una competenza straordinaria; il Parlamento è una risorsa straordinaria, e lo dico davvero rivolgendomi a tutte le forze politiche. Io qui, da cittadino entrato in quest'Aula quasi a digiuno di politica, ho avuto modo di conoscere persone di grande esperienza politica e professionale. Non è forse meglio rischiare di tornare alla propria vita piuttosto che continuare ad alimentare, sostenere, difendere e garantire lo stato di ordinaria amministrazione in cui versa questa maggioranza? Abbiate coraggio, abbiate coraggio, perché oggi ognuno di noi deve ricordare di portare sulle proprie spalle la responsabilità del futuro di questo Paese.

L'unico stato di emergenza che questo Paese ha in questo momento, a mio e a nostro avviso, è la permanenza di questo Governo. *(Applausi).* dovremmo pensare un po' più a questa situazione; sarebbe meglio che ci soffermassimo sul punto. È la permanenza di un Governo che ha approfittato di un momento così tragico, così difficile, per compiere azioni di forza sistematiche e continuative per imporre, attraverso l'istituto dei decreti-legge e gli abusi della fiducia chiesti a un Parlamento completamente esautorato, il completo imbavagliamento del Parlamento stesso, che è la voce dei cittadini. Noi stiamo consentendo - dico noi, ma guardo dall'altra parte dell'emiciclo - la morte della democrazia in modo molle, in modo *soft*, pian piano, quasi senza che la gente se ne accorga; anzi, addirittura con la complicità, perché si parla alla pancia in maniera dissennata, semplicemente perché in questo modo si fanno reagire i cittadini. Ci sono cittadini che pensano, rispetto alle informazioni che sono state date,

la bruttissima comunicazione e la bruttissima immagine che è stata data, quella di un Parlamento inutile, è una grandissima responsabilità per il Parlamento stesso e per la tenuta dell'istituzione democratica, ma tant'è. Noi cercheremo sempre e in ogni modo di ribaltare la situazione e far sì che la competenza, il merito e la corretta informazione escano da queste Aule.

di quelli eletti dalla sera alla mattina, senza un minimo di preparazione, impegno e competenza, anche dieci forse sarebbero troppi. Il Governo ha gestito l'emergenza pandemica in modo del tutto autoreferenziale, stravolgendo i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e della gerarchia delle fonti del diritto, consolidando una prassi che si colloca in netto contrasto con i principi sanciti dall'articolo 70 della Costituzione, che attribuisce proprio al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa. Chi meglio dei parlamentari, infatti, che rappresentano ognuno

portando via le mascherine alle aziende di produzione del territorio, facendole arrivare a Roma e poi non rimandandole più, o a come sta gestendo in questo momento

di dolore dei dirigenti scolastici provinciali - che io chiamo ancora provveditori - che dicono di aver dovuto svuotare le classi di banchi nuovi che avevano perché erano rettangolari;

Questo Governo sta spendendo e sperperando talmente tanti soldi pubblici in azioni inutili che non possiamo non denunciarlo: si comprano i banchi nuovi e intanto non si stabilizzano i docenti, non ci sono gli insegnanti di sostegno e i ragazzini disabili rimangono a casa. di questo Governo dovrebbe provare a vivere nella vita reale, dovrebbe provare a mettersi nei panni di una mamma di un ragazzino autistico che il primo giorno di scuola si era preparato con lo zainetto sulle spalle, pronto ad uscire, arriva a scuola e gli dicono che non può entrare perché non c'è l'insegnante di sostegno e non c'è l'assistente educatore. Oppure, qualcuno dovrebbe mettersi nei panni di quei ragazzi che vengono controllati prima di entrare a scuola, con il distanziamento e i banchi per gli "autoscontri", però dopo si ammassano e si accalcano all'interno degli autobus, perché questo Governo, che ha i paletti ideologici e le fette di salame sugli occhi, non vuole fare le convenzioni con il trasporto privato per aumentare il numero delle corse e fa accalcare i ragazzi o li fa entrare in tre o quattro turni, comunque accalcati. C'è qualcosa di profondamente sbagliato. Questo è un Governo che aveva già dimostrato di non riuscire a governare con le leggi ordinarie; figuriamoci con le leggi speciali e quando dico «leggi speciali» evoco periodi non certo luminosi. *(Applausi)*. Quindi, attenzione, perché la nostra preoccupazione principale è la salvaguardia della democrazia che noi riteniamo veramente in pericolo. Abbiamo cercato sempre di spiegare, anche sulla questione del *referendum*, che un taglio chirurgico di uno solo dei tre poteri dello Stato che hanno bisogno necessariamente di equilibrio per garantire lo Stato di diritto, mette in pericolo la tenuta della democrazia stessa. nel momento in cui andiamo ad azzoppare il Parlamento che è la voce dei cittadini, rendiamo più forte l'Esecutivo e la magistratura. Rendere più forte un Esecutivo che ha già esautorato il Parlamento è estremamente pericoloso. Non mi dilungo perché le questioni sul campo e la cattiva gestione dell'emergenza le vediamo su tutti i giornali: l'economia sta andando a rotoli. l'economia sta andando a rotoli. Non ascoltate la voce degli imprenditori, non ascoltate la voce dei datori di lavoro, non avete voluto introdurre i *voucher*, non avete voluto creare un semestre bianco che sollevasse un po' dal

siamo anche noi assistenzialisti perché vogliamo dare fondi e risorse alle imprese, alle attività produttive, e ai commercianti. Ma

vuol dire fare in modo che un'azienda, un negozio o un'attività non chiuda e, di conseguenza, che i lavoratori continuino a lavorare e gli gli imprenditori, i commercianti e chiunque altro possano pagare le tasse al Governo. L'assistenzialismo è un'altra cosa. Il Governo si sta comportando come se il Paese Paese avesse sete perché l'acquedotto non funziona e invece di riparare l'acquedotto desse un bicchiere d'acqua a ciascuno per un giorno: il giorno dopo tutti muoiono di sete. Chiudo come ho cominciato: l'unico stato di emergenza per per il Paese è la permanenza di questo Governo. Noi lotteremo fino all'ultimo respiro perché andiate a casa a fare qualcos'altro.

intervengo in merito alla modifica introdotta con il decreto al nostro esame alla legge n. 124 del 2007, relativa al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nella parte relativa alla nomina del direttore dell'agenzia del nostro comparto di *intelligence*. Una vera forzatura, un *blitz* operato dal Governo con decreto. Per la Lega, in tempo di emergenza Covid era comprensibile la necessità di una proroga dei vertici delle agenzie in scadenza al fine di garantire la continuità nella gestione operativa del comparto che, sappiamo, soprattutto nei periodi tra marzo e giugno ha impegnato - e molto donne e uomini che vi operano anche sul fronte del difficile reperimento di dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature sanitarie. Per la Lega, lo sottolineo, è assolutamente chiaro che la responsabilità dei Servizi è in capo al Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, il quale, attraverso gli incarichi fiduciari, nomina i vertici del DIS e le agenzie interna AISI ed esterna AISE. Così come ci è assolutamente chiaro che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha il potere di nominare l'autorità delegata, facoltà cui però il *premier* Conte non ha mai ricorso e secondo la Lega sbagliando. Questi poteri, però, il Presidente del Consiglio dei ministri li deve esercitare nell'ambito di un perimetro chiaro, di una cornice definita che è la legge di riferimento che disciplina il comparto *intelligence* che, lo sottolineo, stabilendo un delicato equilibrio di poteri, è frutto di mesi e mesi di condiviso lavoro parlamentare, di serrati confronti tra le allora forze di maggioranza e di opposizione, lavoro che ha portato a stabilire, per esempio, che il Presidente del Copasir è eletto tra i componenti del Comitato appartenenti all'opposizione. Ed è per questo - e il nostro ragionamento prescinde dalle persone che oggi sono i vertici delle Agenzie, a cui va la nostra la nostra stima e il ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo - che la modifica operata con decreto-legge sulla legge n. 124 del 2007 è profondamente sbagliata nel metodo e nel merito.

è abortito per il rilievi della Corte dei conti, allora per intervenire sulla norma primaria sarebbe stato opportuno ricorrere ad una norma transitoria quante ne abbiamo registrate in questi mesi, per esempio sui vertici delle *Authority*? - e non attraverso la decretazione di urgenza direttamente modificando la legge n. 124 del 2007, senza peraltro un'informazione preliminare al Parlamento anche attraverso le sue articolazioni. Ricordiamo invece tutti che di questo decreto sulla proroga dell'emergenza Covid eravamo stati preventivamente informati dei contenuti - ci fu anche una comunicazione in quest'Aula con tanto di risoluzione - tranne che di questa piccola, particolare, ma assai pesante modifica. Anche il comunicato stampa di Palazzo Chigi all'emanazione del decreto non ne faceva menzione. Perché la modifica della legge n. 124 è sbagliata nel merito? Mentre alla Lega sta bene aver rimarcato che il periodo relativo al rinnovo può essere massimo di quattro anni, confermando l'orientamento originale della legge, quello che non ci piace affatto e che riteniamo assolutamente inopportuno è che questi rinnovi - ripeto, sempre nell'arco massimo di quattro anni - possono avvenire per successivi provvedimenti senza precisarne un numero limite. vuol dire che il Presidente del Consiglio potrebbe rinnovare i vertici ogni sei mesi, addirittura ogni tre mesi, persino ogni mese. Potete capire tutti, onorevoli colleghi, che tutto questo non è funzionale all'indispensabile autonomia dei direttori delle Agenzie. Agenzie. Quale serenità ad operare può avere il direttore di un'Agenzia rinnovato per soli sei mesi o perfino per soli tre mesi? Quale pianificazione e programmazione potrebbe fare, assolutamente indispensabili visti gli scenari geopolitici, in tema anche di economia e di energia, in continuo mutamento? Quale credibilità potrebbe avere il direttore della nostra Agenzia esterna, se rinnovato per pochi mesi, di fronte a un omologo estero, ad esempio il direttore del Mossad israeliano, della CIA statunitense, del MI6 inglese, della BND tedesca, della DGSE francese oppure della SVR russa? SVR russa? Per questo la Lega ritiene necessario intervenire per modificare la norma. Riteniamo opportuno fissare un numero massimo di rinnovi (due, al massimo tre) ovvero, con un ragionamento speculare, fissare una durata minima del rinnovo al fine di garantire uno spazio temporale adeguato di operatività. Per un'auspicata modifica in via parlamentare - lo segnalo - di questa norma sulla nomina dei vertici dei Servizi si sono espressi - lo abbiamo letto ieri dalle agenzie - anche i componenti del Copasir al termine di un'audizione del *premier* Conte, durante la quale si sono svolte e condivise alcune considerazioni. L'auspicio è che la modifica possa intervenire presto in uno spirito di collaborazione, assolutamente indispensabile in un ambito così delicato, rilevante e significativo per il Paese, quale è la sicurezza nazionale della Repubblica. signor Presidente, per dire che la Lega, per la trattazione in Aula di questo provvedimento, ha presentato in tema vari emendamenti, uno anche soppressivo. Se il Governo rinunciasse oggi alla preannunciata fiducia, il Gruppo della Lega sarebbe disponibile a ritirare tutti gli emendamenti tranne l'1.24 (testo 2) che, fissando fino a tre il numero di successivi provvedimenti di rinnovo, sarebbe funzionale a risolvere il problema. Diversamente, se il Governo dovesse confermare la fiducia sul provvedimento, sarebbe sicuramente apprezzabile che il rappresentante dell'Esecutivo oggi presente potesse intervenire per assicurare la disponibilità del Governo a convergere su una prossima proposta parlamentare. Lo sottolineo: il ritocco della norma è assolutamente indispensabile, non solo per i motivi che ho detto in precedenza, ma anche per portare la giusta serenità all'interno del comparto, dove donne e uomini competenti, che dimostrano alta professionalità e spirito di dedizione verso le istituzioni del Paese, vogliono esclusivamente lavorare in serenità ed evitare che il proprio comparto sia continuamente oggetto di attenzioni e di strumentalizzazioni.

Signor Presidente, signori senatori, siamo oggi chiamati a votare la conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2020, recante la proroga dello stato di emergenza, dovuto alla pandemia da Covid-19. Siamo in realtà chiamati a confermare le scelte, che abbiamo assunto ad inizio anno, quando ci siamo trovati di fronte ad una sfida nuova e difficile, con la quale mai avevamo avuto modo di confrontarci. Il Governo ci chiede oggi di continuare a seguire un percorso tracciato con chiarezza, prorogando le misure eccezionali fino al 15 ottobre, che assicurano strumenti di prevenzione e gestione dell'emergenza. Tale emergenza purtroppo è ancora attuale. I dati che registrano aumenti dei contagi non devono spaventarci, ma non possono coglierci impreparati. Siamo stati tra i primi in Europa ad affrontare la pandemia e siamo stati i primi a strutturare in tempi strettissimi una strategia che ha dato i suoi frutti. Non possiamo pensare di sprecare un lavoro ben fatto, perché i dati parlano chiaro e la stessa comunità internazionale lo riconosce: il Governo ha agito con tempismo e ha adottato le misure indispensabili per fronteggiare le nuove difficoltà. e competenza nella gestione dell'emergenza. I numeri che costantemente ci aggiornano sui contagi, nel mondo e in Italia, non sono altrettanto rassicuranti e ci chiamano a prendere coscienza del che l'emergenza è tutt'altro che finita. In questo scenario, la proroga dello stato di emergenza e delle misure conseguenti si pone come indispensabile per fronteggiare la pandemia. Garantire, attraverso la proroga, la continuità dell'azione di contrasto vuol dire avere gli strumenti per non lasciare al virus margini di diffusione, isolando i focolai all'origine e monitorando i contagi. Ciò significa quindi assicurarsi che gli ospedali abbiano personale e mezzi sufficienti, per poter sostenere improvvisi picchi di domanda di assistenza. Quelle che proroghiamo oggi, fino al 15 ottobre, sono tutte le misure che ci hanno permesso di uscire dalla situazione dalla situazione critica in cui ci siamo trovati nei primi mesi dell'anno e che, sono convinta, ci permetteranno di gestire i prossimi mesi. Signor Presidente, è importante ricordare che quanto stiamo affrontando è una sfida che coinvolge il mondo intero, in modo grave e pericoloso. Non possiamo correre il rischio di sottovalutare questo pericolo, né possiamo condividere atteggiamenti troppo permissivi, in contrasto con le dinamiche di assoluta attenzione, che questo subdolo virus impone, né tantomeno possiamo tollerare o avallare atteggiamenti di mero allarmismo. Non possiamo non confermare la scelta della responsabilità e della presa di coscienza del pericolo e sono convinta, in questo senso, che sia indispensabile confermare i poteri affidati temporaneamente ai sindaci e alle autorità sanitarie locali, poter limitare la circolazione delle persone che risultano infette, vietarne l'allontanamento e imporre un periodo di quarantena a coloro che sono venuti a contatto con soggetti infetti. Sono scelte che vanno prese in tempi stretti e con assunzione di responsabilità, nella cornice dell'adeguatezza e della proporzionalità. L'elenco esaustivo di tali strumenti, richiamati nelle norme, attiene a quelle misure che, nei momenti peggiori, hanno fatto la differenza che tuttora fanno la differenza, quando si presenta la necessità di isolare un focolaio, di bloccarne i contagi e di monitorarne gli sviluppi. Sono misure che gli altri Paesi si trovano oggi costretti a prendere, con mesi di ritardo e con effetti catastrofici per la salute dei cittadini. I numeri non mentono: se l'aumento ancora contenuto in Italia ci tiene tutti con il fiato sospeso, i dati riportati in Francia, in Gran Bretagna o in Belgio non lasciano spazio alle chiacchiere. Il numero dei morti negli Stati Uniti non può non suonare come un monito a non abbassare la guardia. Dobbiamo guardare in faccia la realtà, senza allarmismi, ma con raziocinio e prospettiva. Non si possono chiudere gli occhi davanti al pericolo, anzi, bisogna mettere a fuoco e aumentare sempre di più la conoscenza del nemico da sconfiggere. Dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni, che hanno saputo guidare il Paese nei momenti più tragici e garantire loro gli strumenti per agire al bisogno. Abbiamo fiducia nel Presidente del Consiglio e nel Governo, che hanno dimostrato prontezza e competenza nel saper scegliere misure adeguatamente proporzionate ai rischi e ai pericoli legati alla diffusione del virus. Abbiamo fiducia in un Esecutivo che ha saputo sfruttare la tecnologia per usarla al servizio delle necessità delle necessità organizzative dovute all'emergenza sanitaria, permettendo, ad esempio, di svolgere riunioni di organi collegiali in videoconferenza, ma anche di mappare i contagi e strutturare un sistema di allerta Covid-19 con la *app* Immuni. Siamo fiduciosi perché abbiamo visto l'impegno degli italiani, che hanno compreso che la tutela di ognuno comporta lo sforzo di tutti. L'obiettivo primario deve rimanere quello di assicurare adeguati e omogenei livelli di assistenza, perché tutti abbiano accesso alle cure e non si debba mai più - dico mai più - più dover scegliere chi poter curare. Le norme che oggi proroghiamo sono indispensabili allo scopo. Concludo sottolineando che convertire in legge il decreto-legge n. 83 e prorogare l'emergenza Covid-19 vuol dire mantenere un metodo costruito anche sugli errori del passato, ma che ha indubbiamente dimostrato di essere funzionale e vincente: è la scelta di un approccio scientifico ad un problema prima di di tutto sanitario, l'iterazione che permette il miglioramento. rappresentante del Governo, colleghi, è chiaro agli occhi di tutti che la situazione che stiamo vivendo è estremamente complessa sotto ogni punto di vista e come Gruppo Lega lo riconosciamo e lo abbiamo sempre riconosciuto. È tuttavia altresì chiaro ai nostri occhi che gli interventi che il Governo si ostina a mettere in campo per fronteggiare le difficoltà continuano a non essere più appropriati e in troppi casi, come in questo, non sembrano essere quelli indicati dalla nostra Carta costituzionale. Signor Presidente, con il mio intervento di oggi vorrei lasciare ai colleghi che mi hanno preceduto e a quelli che seguiranno l'esame analitico dei contenuti del decreto che ci accingiamo a votare, con le sue problematiche e le sue zone d'ombra, concentrandomi principalmente su come questo decreto e la consequenziale proroga dello stato di emergenza stanno incidendo sul ruolo che in questa legislatura il Parlamento è tristemente costretto a ricoprire. tal fine mi permetto di fare miei e di condividere il pensiero e i concetti espressi in un recente articolo da un giurista e accademico italiano, nonché giudice emerito della Corte costituzionale, il professor Sabino Cassese. Dopo due anni e mezzo di legislatura e pochi giorni dopo il voto per il *referendum* sul taglio dei parlamentari, che per molti mesi ha tenuto banco, è utile tracciare un primo bilancio e chiederci se, dati alla mano, stiamo davvero rispettando il ruolo del Parlamento o se forse è il caso di fermarsi e lavorare per restituire la giusta dignità all'istituzione della quale tutti noi ci onoriamo di far parte. Come sappiamo, il Parlamento è o dovrebbe essere, prima di ogni altra cosa, un organo legislativo, eppure i numeri ci dicono che in questa prima parte di legislatura solo un quarto delle leggi è di iniziativa parlamentare e che è molto elevato il numero dei decreti-legge (ben 63), per un terzo dei quali il Governo ha sentito la necessità di porre la la fiducia in fase di conversione, i consequenziali voti di fiducia, si sono sensibilmente accentuate ed è anche alla luce di ciò che la proroga dello stato di emergenza, che essenzialmente concede al Governo e al Presidente del Consiglio pieni poteri, limitando di fatto il ruolo del Parlamento a quello di semplice passacarte, non può e non deve trovare i favori di chi, come noi, ha a cuore il rispetto della Costituzione e degli organi della Repubblica. Se è vero che in una fase di conclamata difficoltà è essenziale che ci sia rapidità nell'approvazione delle leggi, spiace dover sottolineare che il Governo non è stato in grado di raccogliere appieno i frutti e i benefici di cui fin qui ha potuto godere. I dati ci dicono che i tempi medi di approvazione delle leggi parlamentari si dimezzano quando parliamo di quelle di iniziativa governativa e ci illustrano in maniera inconfutabile come, specie nell'ultimo periodo, il ruolo del Parlamento sia dovuto necessariamente mutare e come lo stesso abbia dimostrato un'inesausta capacità trasformativa, così come la definisce appunto il «Rapporto sulla legislazione» del 2020. Le migliaia di emendamenti che sono andati a modificare sostanzialmente i vari decreti-legge che si sono succeduti negli ultimi mesi danno l'idea chiara di un Parlamento sempre meno indipendente e sempre più a rimorchio del Governo, che non legifera, ma emenda, e che si condanna a un ruolo interstiziale, con l'insoddisfacente risultato di tante leggi e poco Parlamento, pochissimo Parlamento. A dispetto di quello che ci si potrebbe attendere, il Parlamento da parte sua non sembra aver dimostrato scarsa voglia o attitudine al lavoro; anzi, tutt'altro. I dati ci parlano di un numero elevatissimo di disegni di legge presentati, di interpellanze, di interrogazioni, di tante indagini conoscitive avviate o svolte e di grande solerzia anche nelle attività di controllo. Vi è dunque, nell'operato del Parlamento, un evidente e ingiustificabile problema di incidenza e di efficacia. Un altro aspetto che a noi è tristemente noto e che il suddetto rapporto sulla legislazione mette in risalto è il fenomeno del monocameralismo alternato: una delle due Camere è di fatto sempre costretta ad approvare, sostanzialmente ad occhi chiusi, il testo trasmesso dall'altra parte per evitare la decadenza dell'atto. Riteniamo sia giunta l'ora di porre fine a queste inique consuetudini, se è a questo che serve la vostra proroga dello stato di emergenza. Se questa è la vostra idea di democrazia e di rispetto delle istituzioni, perdonateci, ma ci troverete sempre e comunque sull'altra sponda, sempre e comunque a difesa dell'Italia, dei suoi valori, dei suoi cittadini e della centralità democratica del Parlamento. Il continuo utilizzo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (questa nuova e a quanto pare indispensabile moda di normare) e la leggerezza con la quale questo Governo e questa maggioranza dimostrano di giocare con i decreti, abrogando le norme di altri decreti-legge in fase di conversione, inserendo proroghe in blocco dei termini di delega in scadenza o tralasciando tutte le deroghe alla legislazione vigente con proroga dell'emergenza, sono l'emblema di una pagina triste, nera e mortificante che state regalando al nostro Parlamento. Pur non condividendo minimamente il vostro *modus operandi*, qualora questo portasse a dei risultati probabilmente, per il bene del nostro Paese, le nostre critiche sarebbero meno pressanti. Ma purtroppo il vostro modo di agire, oltre a non essere in linea con i dettami delle nostre istituzioni, porta solo a un caos per nulla organizzato; e a farne le spese sono, come sempre, i cittadini italiani, che si ritrovano con leggi frammentari e incomprensibili e mai davvero risolutive. Come tutti noi ben sappiamo - anche se alcuni probabilmente fanno talvolta finta di non ricordarselo - tutta questa massa di norme richiede ulteriori precetti applicativi e a oggi il Governo si ritrova con circa 300 decreti attuativi da emanare; non ci si accorge - o forse sì che chi pensa di agire in questo modo convinto di abbreviare i tempi in realtà non fa altro che produrre distorsioni e vincoli, che rendono ancora più difficoltosa la vita dei cittadini, le uniche vere vittime dell'operato di questo Governo. Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, voglio dirle che, esaminando il decreto-legge oggi in discussione, menzione approfondita meriterebbe - come già fatto dal collega senatore Arrigoni - ciò che è accaduto alla Camera dei deputati sul tema della proroga dei vertici del DIS, dell'AISE Molto si è detto e molto altro sarebbe interessante poter dire, ma il tempo è tiranno e su questo mi limito a rimarcare che il Governo e la maggioranza che lo sostiene si sono resi protagonisti di un'ennesima bruttissima figura, dimenticando che in passato l'opacità della gestione di questi apparati statali ha dato adito a diversi episodi dubbi che si trascinano ancora oggi. C'è poi almeno un'ulteriore inspiegabile mancanza nel decreto in esame, che riguarda la necessità di conferire tutela ai cosiddetti lavoratori fragili, una categoria che l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge cura Italia aveva protetto, stabilendo che l'assenza dal lavoro per portatori di disabilità e affetti da gravi patologie fosse equiparata al ricovero ospedaliero. Tale tutela era stata poi prorogata dal successivo decreto rilancio fino al 31 luglio 2020, ma poi è scomparsa nei successivi provvedimenti e non è stata fatta rientrare tra le altre proroghe previste fino al 15 ottobre 2020. Oggi migliaia di lavoratori fragili si sono ritrovati davanti alla scelta di rientrare comunque in servizio, con tutti i rischi del caso, oppure restare a casa utilizzando ferie o malattia tramite certificato medico, con il rischio di superare il periodo di comporto, che consente al datore di lavoro di procedere con il licenziamento. Se c'era una disposizione che andava effettivamente prorogata con il decreto-legge in commento era proprio questa. Da qui si doveva partire, dalla tutela dei maggiormente bisognosi, e invece su questo punto non è stato fatto inspiegabilmente nulla, tranne correre ai ripari in Commissione con un ordine del giorno. Il Governo, però, a essere onesti, una cosa l'ha fatta, la stessa cosa che fa da sempre. Ha prima invocato l'emergenza, quando si è trattato di richiedere i pieni poteri, e poi se n'è dimenticato completamente quando è arrivato il momento di tutelare i soggetti più deboli, quando è arrivato il momento di tutelare i cittadini italiani.

non riteniamo che debbano essere mantenute delle precauzioni, che vanno osservate per prevenire la diffusione del virus,

proseguire con le misure di sicurezza, che vanno semmai ragionate e discusse, seriamente e apertamente, con gli esperti e con la comunità scientifica.

Ci siamo opposti, perché in questi mesi lo Stato d'emergenza è stato usato dal Governo per scopi che non hanno nulla a che fare con l'epidemia e, comunque, e, comunque, in modi ampiamente scorretti, a cominciare dall'uso del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di ciò che la Costituzione prevede si possa usare in casi di straordinaria necessità ed urgenza. questi casi di straordinaria necessità ed urgenza, che determinano l'uso del decreto-legge, sono stati ampiamente abusati nel passato, si è ritenuto che il sistema alla faccia della Costituzione e alla faccia dei Padri costituenti, che di emergenza se ne intendevano, essendo appena usciti da una guerra che aveva fatto centinaia di migliaia di morti (una guerra tra italiani, anche in Italia, con l'occupazione straniera,

il Presidente della Repubblica non può e non ha necessità di apporre la sua autorizzazione, come per i decreti-legge, che non viene necessariamente annunciato alle Camere

che, nel momento dell'emergenza, quando hanno cominciato a fioccare questi decreti del Presidente del Consiglio, noi non abbiamo denunciato questo grave problema per senso di responsabilità. In una situazione in cui c'erano centinaia di morti al giorno, non abbiamo voluto dare l'impressione di disunirci su un punto che sarebbe stato difficilmente percepibile, specialmente in una informazione monopolizzata dal Presidente del Consiglio, che compariva nelle ore di massimo ascolto per fare comunicazioni che avrebbe dovuto fare in Parlamento, non scegliendo scegliendo l'ora del massimo ascolto con la consulenza di Casalino (che, giustamente, è pagato molto più di un parlamentare e, pertanto, ha un ruolo molto più importante). Non abbiamo fatto polemica all'epoca ma adesso, con la situazione che è cambiata, dobbiamo denunciare questo fatto: è stata violata la Costituzione sulla questione dell'urgenza con il pretesto dell'urgenza. L'urgenza c'era,

È stata violata la Costituzione anche dal punto di vista dell'estraneità di materia. Lì la lettera del Presidente della Repubblica si riferiva a un argomento, ma ce ne sono ben altri di argomenti. Faccio riferimento, per esempio, alla decreto rilancio grazie alla quale, per pura casualità, il padre della compagna del Presidente del Consiglio si è trovato, da un giorno all'altro,

Mi viene ora in mente una cosa. Quando è stato approvato il decreto-legge (che è firmato dal presidente del Consiglio Conte e da un altro Ministro), il Presidente del Consiglio è uscito dalla sala del Consiglio dei ministri, oppure lo ha approvato?

è stata usata anche per i banchi. L'ottima collega Gallone ha parlato del problema funzionale dei banchi, che non ripeto perché non si può dire meglio di come lo ha illustrato lei.

per fare profitto su banchi verosimilmente acquistati presso il Paese di riferimento della politica estera di questo Governo, ossia la Repubblica popolare comunista cinese, alla quale si fa anche riferimento come modello di democrazia e magari la si fa entrare nel nostro sistema informativo e di sicurezza. *(Applausi)*. Come è stato detto dal senatore Arrigoni, inserita anche una previsione che grida vendetta, ovvero la proroga dei servizi di informazione, che mette nelle mani del Presidente del Consiglio la minaccia giornaliera, rispetto ai servizi di informazione, di poterne rimuovere i capi. In altre parole, questi devono obbedire e fare gli interessi

il Parlamento vigila sulle leggi da approvare e deve approvarle a viso aperto e non con la fiducia, come si farà anche oggi, nonostante ci siano soltanto 29 emendamenti. *(Applausi)*. La fiducia costringe

grandissime e gravissime. Noi ci batteremo per difendere la democrazia e il Parlamento fino all'ultimo respiro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretari, mi spiace che oggi il ministro Speranza non sia in Aula: avrei voluto rivolgermi direttamente a lui per dirgli che ogni volta che si rapporta con il Parlamento lo fa con apparenti disponibilità e affabilità, ma in realtà leggendo il suo comportamento si possono intravedere l'arroganza e il disprezzo per qualunque contributo possa arrivare da questo Parlamento, tant'è che ha sempre respinto qualsiasi soluzione e rigettato ogni azione, anche se di buonsenso, proposta dalla minoranza. Sapete chi mi ricorda? Il marchese del Grillo, quando con il suo sorriso *snob* si atteggiava rispetto alla gente ritenuta inferiore, e vi risparmio la citazione. Questo provvedimento di proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 dimostra chiaramente il vostro atteggiamento carico di arroganza e disprezzo per le persone meno privilegiate di voi. Davvero pensate che gli italiani vi credano ancora sulla necessità di prorogare lo stato di emergenza? State andando avanti a stati di emergenza dal 31 gennaio 2020. È una vergogna.

Ormai siete allenati nel violare a vostro piacimento i diritti costituzionalmente garantiti, come avete fatto con il *lockdown* su tutto il territorio nazionale, esautorando il Parlamento dalle sue prerogative. Da mesi state impedendo ai rappresentanti del popolo di esercitare le loro funzioni, che - ripeto - sono costituzionalmente garantite, sperando che qualcuno mi ascolti. State nascondendo la verità, ovvero che non c'è oggi alcuno stato di emergenza, ma solo la vostra manifesta incapacità. Vergognatevi. Potete raccontare al mondo che avete vinto alle ultime elezioni, ma la realtà è che la vostra emorragia di consensi è inarrestabile. Dov'è la vostra onestà morale? Gli italiani non vi vogliono più, ma voi continuate sadicamente ad imporre la vostra presenza e intanto - lo dico soprattutto ai parlamentari del Gruppo MoVimento 5 Stelle - dilapidate i vostri voti facendovi lentamente cannibalizzare dal PD, ben più scafato di voi incapaci. Che triste epilogo il vostro! Volete vedere gli italiani con il cappello in mano in attesa dei vostri *bonus*, vero? Ma vi sbagliate. Gli italiani hanno molta più dignità di quanto pensiate. Gli italiani vogliono un Governo all'altezza di un nuovo patto con lo Stato, che preveda l'abbattimento del cuneo fiscale per tutti, per aiutare finalmente le aziende senza che scappino all'estero per la pressione fiscale; un patto per evitare che le partite IVA si estinguano; un patto per i lavoratori che non potrete tenere per sempre in cassa integrazione, per i pensionati che non arrivano a fine mese. Dovete vergognarvi. Dopo otto mesi lo avete un piano pandemico? Quale idea di sanità avete? Dov'è che collocate l'individuo nella vostra visione della sanità? In tutti i provvedimenti parcellizzati che mettete in campo per sistemare gli amici vi siete dimenticati delle persone. È chiedere troppo dare il proprio contributo per una sanità che metta al centro il paziente? Siete qui a chiedere una proroga dello stato di emergenza, ma perché invece non avete lavorato ad un piano organico e strutturato? Vi rendete conto del disastro che state facendo nella scuola, con un Ministro che dopo sette mesi è riuscito a far iniziare le scuole senza insegnanti, ma con i banchi a rotelle che permettono ai ragazzi di correre per i corridoi e di giocare agli autoscontri

per se stessa sicuramente, dal momento che andrete a casa, ma chi pagherà il danno arrecato ai nostri figli? Dovete pagare voi! Invece di venire in quest'Aula a chiedere proroghe, dovete dire a questo Parlamento e agli italiani quale futuro immaginate per i nostri figli. È difficile pensare a concorsi regionalizzati per dare risposte agli studenti, alle famiglie agli insegnanti sulla base del fabbisogno reale? Perché non mettete lo studente al centro? Serve urgentemente un sistema di valutazione della formazione e del percorso scolastico, compreso quello degli insegnanti. Gli studenti vengono formati per il mondo del lavoro se gli insegnanti sono di qualità, con competenze misurabili; invece state distruggendo la ricerca e i ricercatori, obbligandoli a scappare all'estero. un danno incalcolabile, che va oltre il buon gusto. Siete davvero spudorati. Ciò che che mi lascia interdetta è l'assordante silenzio del Presidente della Repubblica: dov'è il garante delle istituzioni e della Costituzione? Dove si trova il Presidente dopo tutti questi mesi?

Per caso il Presidente della Repubblica ha perso l'uso della parola? Abbiamo bisogno di un suo intervento urgente conclusione, avrete anche la compiacenza delle altre istituzioni, ma la certezza è che non avete il popolo con voi e quando questa farsa finirà, voi andrete a casa e il Centrodestra tornerà a governare nell'interesse dei nostri concittadini e non delle *lobby* che state disperatamente cercando di inculcare nelle stanze delle nostre istituzioni

di devastante conflittualità politica, che continua anche oggi su un provvedimento di questa natura, appare incomprensibile ed eccessivo. Parlare di questo come di un provvedimento che mina l'ordine democratico del nostro Paese appare una polemica ormai stucchevole oltre che strumentale: stucchevole perché va avanti ormai da troppi mesi, come se le scelte del Governo fossero state dettate

una recrudescenza del virus, con dati - proprio ieri li pubblicava l'Organizzazione mondiale della sanità - che mettono in evidenza che si sono raggiunti i due milioni di contagi

per rimanere ai Paesi europei più vicini. Non credo ci sia stato un eccesso dal punto di vista del Governo: credo si sia preso atto di una situazione complicata. Noi di Italia Viva siamo stati anche i più critici in alcuni momenti rispetto alla proroga dello stato di emergenza. Ricordo che in Senato parlammo del fatto che bisognava comunque fare talune valutazioni prima di arrivare a una proroga eccessivamente lunga. Ma, alla luce di quanto sta accadendo, mi sembra sia sia stato giusto aver pensato a un provvedimento di questa natura, che tra l'altro ha un contenuto meramente tecnico. Si tratta sostanzialmente di fornire gli strumenti

19 del 2020, ovvero quello che ha costituito la cornice giuridica entro la quale collocare i DPCM e le ordinanze del Ministero della salute. In quel decreto-legge sono indicati tutti i possibili campi di intervento, che sono quelli che hanno caratterizzato gli ultimi mesi di vita, le chiusure,

questo può aprire un altro fronte di polemica e considerazioni politiche, ma così è stato. Si ridà equilibrio al rapporto tra Stato e Regioni. Inoltre, il decreto-legge non ha niente di scandaloso.

che consentiranno a questo Paese di avere più tempo rispetto ad alcuni settori importanti di governo dell'emergenza sanitaria. In quell'allegato sono infatti contenute proroghe relative alla possibilità di assumere personale specializzando nel campo della medicina o personale

Penso poi anche allo *smart working* per chi è in condizioni di disabilità, un elemento introdotto nell'esame della Camera, così come all'estensione a novanta giorni dei piani terapeutici, che rappresentano un importante supporto

come dovrebbe essere visto. Mi pare che il quadro politico abbia espresso anche questo. Crediamo che questo sia un provvedimento che vada licenziato anche con una certa celerità, perché - se ricordiamo bene - la proroga dello stato di emergenza è stata comunicata a questo ramo del Parlamento il 28 luglio; i tempi sono sono trascorsi e il provvedimento deve vedere la sua conversione per chiudere anche questa ulteriore fase. siamo anche noi convinti che questo è un Paese in difficoltà dal punto di vista economico. È stato messo in campo un ventaglio di provvedimenti anche dal punto di vista dell'impegno economico-finanziario non irrilevante.

e deve consentire al Governo di avere gli strumenti per mettere celermente in campo quello che serve per fronteggiare

il livello di complessità del problema Covid dal punto di vista mondiale è tale per cui dovremmo cercare di sottrarre il dibattito dalla polemica politica continua e vedere oggettivamente le cose di cui

Signor Presidente, colleghi senatori, Ministri e Sottosegretari presenti, la prima cosa che mi viene da dire rispetto a tutto quello che si sta discutendo è che con la salute non si scherza.

lo abbiamo già visto. Peraltro, possiamo ancora permetterci di parlarne e di decidere come affrontare e migliorare determinate situazioni, perché lo stiamo controllando. Guardate solo all'apertura delle scuole: al di là di tutte le criticità che possono essere emerse, anche l'apertura delle scuole ci ha dato un grande risultato perché il virus è stato tenuto sotto controllo.

del Parlamento - come è stato detto molto bene prima dai miei colleghi - come aver dato la possibilità di assumere specializzandi, di aver aggiunto nuovi posti letto nelle terapie intensive, aver implementato le cosiddette USCA, cioè le unità speciali di continuità assistenziale

Bisogna anche cercare di capire che era essenziale farlo, perché il nostro Paese, attraverso la scuola e l'educazione, può fare passi grandi, perché il futuro viene da quei ragazzi che oggi vanno a scuola in maniera diligente. Credo che questo sia davvero un passaggio importante che noi dobbiamo fare,

Grazie

delle posizioni fra gli schieramenti vada riletta guardando quella mozione. Non è una litania - mi dispiace che non sia presente il collega Grimani, ma vi prego di riferirglielo, come anche alla collega Boldrini - il fatto che si dica che c'è un problema di limitazione delle libertà, né è una contrapposizione strumentale. Il centrodestra aveva fatto una richiesta precisa - e alcuni colleghi della Lega nei loro interventi lo hanno ricordato - ossia che al Parlamento fosse portato un piano nazionale di sorveglianza epidemiologica

Pone invece questo problema, che riguarda parecchi articoli della Costituzione (ovvero il 13, il 16, il 17, il 18 e il 19) e le libertà fondamentali dei cittadini, per il semplice motivo che tali libertà sono state compresse, perché il nostro Sistema sanitario non era pronto ad affrontare il numero dei malati e l'emergenza. Abbiamo tenuto un Paese siamo stati chiusi, perché non c'era un Sistema sanitario in grado di reggere quell'onda d'urto. siamo in grado di reggere l'onda d'urto, se ritorna, in modo tale da non limitare le libertà fondamentali dei cittadini. Quando chiediamo il piano epidemiologico; quando chiediamo informazioni sulla questione dei vaccini antinfluenzali; quando chiediamo a che punto è lo stato dell'arte con riferimento alle strutture sanitarie, la domanda che c'è dietro è

a non chiudere la gente in casa e a riavere un Sistema sanitario che regge? Se a questa domanda non viene data una risposta, significa che lo stato di emergenza, così come richiesto fino al 15 ottobre - nella speranza che il presidente Conte non torni a chiedere una proroga fino al 31 dicembre non è giustificato in rapporto alle libertà fondamentali dei cittadini. E, quindi, hanno ragione i costituzionalisti quando ci dicono che siamo fuori dalla Costituzione, perché i limiti delle libertà fondamentali devono essere basati non sul timore di un evento, ma sulla legge, tenuto conto che l'evento si è verificato. Aggiungo che,

un concorso colposo dello Stato, cioè il concorso colposo di un Governo che - a nostro avviso - non ha approntato tutto ciò che era necessario. Abbiamo avuto degli avvisi da questo punto di vista: lo abbiamo visto per la scuola

Avendo capito che la pandemia non è più un'ipotesi astratta di scuola, ma è un qualcosa che può comunque colpire - sia che venga causata da questo o da altri virus - il punto sostanziale è che dobbiamo essere pronti ad affrontare

della maggioranza, perché significa procedere a scatola chiusa, senza sapere esattamente quale sia la strada e, soprattutto, cosa si sia costruito in questi mesi per non

di un argomento che può essere tranquillamente affrontato in via ordinaria, attraverso una votazione in Parlamento, senza che vi sia - lo dico in maniera precisa - la forte e arrogante imposizione della questione di fiducia. Perché continuare con questo meccanismo che sta sostanzialmente esautorando

veloci, che non si impastassero con la burocrazia e tutto il resto. *Ex post* possiamo dire che avete detto una grande bugia perché è oggettivo che, per come è partito, l'anno scolastico tutto è tranne che ordinato, gestito con i giusti tempi

Questo non va bene ed è veramente grave che tutto ciò avvenga in una situazione di pericolo e di crisi per la salute dei cittadini, perché di questo stiamo parlando. Dopodiché, qui dentro ci sono da fare delle considerazioni, signor Presidente.

per costruirsi un sistema di potere autoreferenziale. Lo dico perché resti agli atti e perché resti a verbale: si sta costruendo un sistema di potere autoreferenziale e lo sta facendo nel peggiore dei modi, utilizzando addirittura meccanismi come la decretazione di urgenza.

statene ben tranquilli - perché finché c'è Covid c'è speranza; sembra un gioco di parole, ma nella realtà del Governo abbiamo capito che purtroppo questa è tutt'altro che una frase fatta. I comitati di esperti, tutte le relazioni del Comitato tecnico-scientifico, gli Stati Generali, eccetera: avete dato l'impressione di avere tutte le soluzioni a portata di mano. Non è ammissibile che si sia arrivati a un decreto che mette in stato di emergenza il Paese ancora con il caos nella scuola. Signor Presidente, negli scorsi giorni mi sono arrivate delle segnalazioni da parte di operatori della scuola e anche di genitori; può succedere in qualsiasi Comune. Sono andato a vedere nelle scuole del mio Comune, nelle scuole superiori di Tradate, dopo aver letto una notizia che mi ha inviato un genitore, il quale scrive: «Ma queste sono le mascherine che avete scelto per i nostri ragazzi? Ma qualcuno le ha provate? A mia figlia sono grandissime, non riesce neanche a vedere, le coprono gli occhi. Come fanno questi ragazzi a tenerle per sei ore? E in più sotto sono aperte, è come non averla. Ma come fate così a proteggere i nostri figli? Non comprendo, mi viene voglia di non mandare i miei figli a scuola». Andiamo a vedere. Signor Presidente, mi sono recato agli istituti superiori di Tradate e ho trovato questi pacchetti che sto mostrando; queste sono le mascherine inviate nelle scuole,

Siamo in Parlamento; lei deve stare dalla parte del Parlamento e non del Governo.

E aggiungo di più: l'inganno che c'è scritto qua sopra, signor Ministro. Qui c'è scritto: «Mascherina chirurgica tipo 1». Sotto c'è scritto piccolo piccolo, con parole che non si leggono se non con la lente d'ingrandimento: «Le maschere di tipo 1 non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o altre attività mediche con requisiti simili». Mascherina chirurgica! Allora, signor Presidente, se questo non è un argomento degno di entrare in Parlamento, cosa ci stiamo a fare noi qua dentro? Questo è quello che sta succedendo nelle nostre scuole. Questo è quello che il Governo ci aveva detto che non sarebbe accaduto: l'approssimazione e, addirittura, far passare una cosa per un'altra. Sono molto preoccupato. E noi abbiamo tutte le ragioni per essere preoccupati, signor Questa non è una situazione normale e, se siamo in stato di emergenza, voi avete messo una persona che si chiama Arcuri a risolvere questi problemi. Questo è quello che sta facendo Arcuri. Questo è quello che non deve succedere e su questo dovete rispondere in Parlamento e ai cittadini.

il 31 maggio il primario del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, ha dichiarato: «Il Covid-19 non esiste più. Qualcuno terrorizza il Paese». Quattro mesi dopo, nel mondo vengono quotidianamente scoperti altri 315.000 nuovi positivi e in Italia più di 1.500. 21 agosto, il *leader* della Lega Matteo Salvini, ha detto: «Ora il Covid-19 è gestibile senza allarmismi. È assurdo parlare di emergenza e mancanza di emergenza. Questo è terrorismo per mantenere il potere». stesse frasi che abbiamo risentito poc'anzi in Aula. Terrorismo è quel che cerca di fare qui la Lega da alcuni anni a questa parte, spaventando gli italiani per racimolare consensi, inventandosi paure che non hanno riscontro - queste sì - da nessun dato ufficiale. Per quanto riguarda il mantenimento del potere, gli italiani con questa tornata elettorale sono stati chiari: il Governo deve andare avanti. E lo hanno comunicato in maniera democratica: altro che colpo di Stato. Sono alcuni mesi che una parte della politica, dell'informazione e dell'opinione pubblica ripete che il Covid-19 non rappresenta più un pericolo, che l'epidemia è passata. A marzo l'Italia era stata investita da un TIR chiamato coronavirus e tutti noi temevamo per il nostro futuro; secondo gli oppositori al Governo, oggi non è più così e il pericolo è scampato. A marzo tutti noi tolleravamo lo stato di emergenza proprio in virtù di quella realtà; oggi molti lo giudicano un'imposizione degna di uno Stato totalitario. Dobbiamo smetterla di essere antiscientifici e con la memoria corta. A marzo nel mondo si contavano meno di 100.000 nuovi casi giornalieri di Covid-19; oggi sono più di tre volte tanto. Il coronavirus sta mietendo vittime ovunque. I contagiati hanno superato quota 31 milioni e i morti stanno per varcare la soglia psicologica di un milione: un milione di vittime che sarebbe stato in buona parte evitabile se i Governi di tanti Paesi avessero preso seriamente la lotta all'epidemia, se avessero avuto il coraggio che ha avuto il Governo italiano. Il nostro Governo ha adottato provvedimenti straordinari di necessità e di urgenza - come stabilito all'articolo 77 della Costituzione - aventi forza di legge, senza penalizzare il ruolo centrale del Parlamento. Ha messo in atto uno strumento efficace rispetto ad una situazione in perenne cambiamento, che richiedeva continui aggiornamenti su regole e azioni da intraprendere; norme da alcuni giudicate restrittive e che, invece, sono a protezione della salute. Tanti, troppi esponenti politici che si trovano in quest'Aula accusano il Governo di aver distrutto l'economia: punti di vista miopi e poco attenti al quadro complessivo. Le previsioni qualche mese fa davano il PIL in calo del 12 per cento. Grazie al comportamento restrittivo del Governo, oggi quegli stessi organismi nazionali e internazionali dicono che la ricchezza prodotta dal Paese diminuirà del 9 Magari alla fine dell'anno l'economia italiana avrà avuto un rimbalzo ancora maggiore rispetto al 3 per cento attuale. Le regole rigide imposte dal Governo grazie all'esistenza dello stato di emergenza permettono all'Italia di avere una ripresa economica migliore rispetto agli altri Paesi europei. Noi ne siamo usciti prima, meglio e soprattutto con minor rischio di una seconda ondata. Pensate al contraccolpo psicologico ed economico che stanno subendo gli imprenditori del Regno Unito in questo momento. E che dire di quelli della Spagna, della Francia, di parte della Germania, del Belgio e dell'Olanda? C'è poi la questione sanitaria. Chi ha una visione miope delle cose giudica le questioni sanitarie come temi che riguardano solamente la salute delle persone, non rendendosi conto che una società sana dal punto di vista medico è anche più florida dal punto di vista economico. Ogni persona che va in ospedale per curarsi rappresenta un costo non da poco per la società. Tenere il Covid lontano dai nostri concittadini vuol dire proteggere la salute e non solo, in quanto significa anche proteggere i conti di questo Paese. Il coronavirus, oggi come non mai, sta circolando in tutto il mondo, mettendo in ginocchio, uno dopo l'altro, decine di Paesi. Il Covid ci ha dimostrato che un'epidemia da coronavirus non conosce confini ed è in grado di spostarsi in meno di ventiquattr'ore da un continente all'altro e di diffondersi all'interno di un piccolo territorio con una velocità sorprendente, che purtroppo abbiamo vissuto sulla pelle di tanti di noi. L'esperienza ci ha insegnato che la rapidità della reazione da parte delle autorità è uno degli elementi chiave per riuscire a contenere il contagio. L'esperienza ci ha anche insegnato che il miglior antidoto al Covid, in attesa della cura, resta il distanziamento sociale, che è garantito da una serie di regole possibili solo grazie all'esistenza dello stato di emergenza. Quando questo cesserà, quelle regole decadranno. Le regole per la gestione del Covid nelle scuole sono possibili solo grazie all'esistenza dello stato di emergenza; la limitazione di spettatori negli spettacoli dal vivo è possibile solo grazie all'esistenza dello stato di emergenza. Lo *smart working* utilizzato in maniera massiccia, la cassa integrazione straordinaria a protezione dei dipendenti di piccole aziende, il divieto di licenziamento, le proroghe alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo per personale medico e infermieristico: sono tutte cose possibili solo grazie all'esistenza dello stato di emergenza. È di questi giorni l'ennesimo elogio da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità al Governo italiano, indicato come il più virtuoso degli Esecutivi in Europa e nel mondo democratico. In Francia i contagi giornalieri hanno superato nuovamente quota 10.000, in Germania quota 2.000, nel Regno Unito 4.000, in Belgio e Olanda, che hanno una popolazione molto inferiore alla nostra, quasi 2.000; Israele è di nuovo in *lockdown.* È vero, lo stato di emergenza non è accettabile in condizioni normali. È vero, lo stato di emergenza è da augurarsi finisca al più presto e resti nei nostri ricordi, sperando che il suo spettro non ritorni più nel futuro. però non sono tempi normali: questo è il tempo della pandemia, questo è il momento di cercare di impedire che lo *tsunami* travolga ancora una volta l'Italia, come sembra sia facendo nei Paesi nostri vicini. È per questo che lo stato di emergenza è necessario e non rappresenta un pericolo, se non per coloro che si nutrono della paura e del fatalismo sconsiderato.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato del Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge n. 1928, di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, nel testo proposto dalla Commissione, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. Sospendo pertanto la seduta in attesa delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che è immediatamente convocata in sala Pannini, in ordine all'organizzazione del dibattito sulla fiducia. *(La seduta, sospesa

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 15,30.

una nuova finestra"). Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà. Signor Presidente, già da metà luglio avevamo avuto modo di rimarcare come, a nostro avviso, non sussistesse alcuna evidente motivazione per prorogare lo stato di emergenza, posto che, contrariamente a inizio pandemia, si erano sviluppate conoscenze e competenze tali da garantire una diversa presa in carico dell'eventuale recrudescenza epidemica, in modo da far sì che i malati non dovessero, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, neppure "avvicinarsi" alle terapie intensive. Ovviamente, avevate altre motivazioni. Una per tutte, la proroga del commissario e anche di quella non si sentiva il bisogno. Ma tant'è! Quello di cui invece c'era bisogno, un vero piano anti pandemico, non lo avete ancora processato. L'ultima chiamata avrebbe potuto - e dovuto - essere il provvedimento in discussione, ma non ve n'è nessuna traccia.

nostre proposizioni e raccomandazioni, incidenti sul decreto in conversione, che avrebbero potuto porre rimedio almeno ad alcune delle gravi mancanze e incongruenze, di cui si accorge il Paese e che voi continuate a ignorare, non prendendo neanche in considerazione, a colpi di fiducia, di adottare le misure selettive adeguate di governo del rischio di quella che è una co-pandemia cronico-infiammatoria ed infettiva al tempo stesso, coniugando la necessità di normalizzazione dei tempi di erogazione delle prestazioni ed interventi per patologie diverse dal Covid-19

con misure emergenziali di protezione delle persone e nei luoghi più a rischio, su cui si deve assolutamente intervenire: anziani, malati e cronici negli ospedali e nelle residenze sanitarie assistenziali e continuare a fare Commissioni aiuta pochissimo. Varrebbe invece la pena di testare, in aggiunta agli ordinari, almeno un milione e mezzo al mese di pazienti a maggior rischio

del tutto eccezionalmente, si poteva ascrivere la necessità di mantenere lo stato emergenziale fino a metà ottobre. Ci siamo disinnamorati a continuare a parlare al vento, è giunto il momento che valutiate di interrompere un'esperienza di Governo che, oltre alle manifeste incompetenze,

e non avete mai dato contezza di ascoltare suggerimenti e proposte che, con il senno di poi, è troppo facile definire appropriate. Siete riusciti nel "capolavoro" di affossare l'economia e state lavorando pervicacemente per rilanciare l'epidemia: forse è troppo! Temiamo che il prolungarsi della vostra permanenza al Governo

a quanto alacremente state ponendo in essere: il dramma vero è che le conseguenze di questa gestione costeranno carissime e si pagheranno nei prossimi trent'anni. Avete bruciato un'opportunità per proiettare il Paese dall'arretratezza burocratica,

che avrebbero dovuto "educare alla responsabilità" anzitutto dello Stato nel mantenere i propri impegni, invece a non onorare le sue obbligazioni, posto che ha debiti verso fornitori per oltre 50 miliardi di euro e non vi è traccia di uno "straccio" di codicillo che ne preveda il suo assolvimento.

istanze che, con la scusa del *lockdown* e dello *smart working*, non vengono neppure prese in considerazione: anche questo non solo non aiuta, ma affossa l'economia reale perché, in un momento di così alta tensione,

di tutta evidenza che ci si trova di fronte a una condizione nella quale non vi dimenticate di non vi dimenticate di chiedere alle imprese e ai cittadini l'assolvimento dei loro obblighi, ma non vi sembra sia ancora giunto il momento di riequilibrare il rapporto tra Stato e cittadini, «io faccio quel che dico, ma tu fai quel che devi». Assistiamo alla rivendicazione degli adempimenti fiscali e all'imposizione delle restrizioni sui comportamenti individuali, ma lo Stato continua a non assolvere ai suoi doveri, incapace di trasformare in un'opportunità di crescita gli investimenti in sanità, con una strategia sanitaria a valenza economica di riqualificazione e autentica prevenzione, realizzabile solo evitando gli sprechi, cosa che continua a non essere fra le priorità di questo Governo. Ci sembra che ce ne sia abbastanza!

in questa sede intervengo, ovviamente, innanzitutto per motivare il no chiaro e limpido del Gruppo Fratelli d'Italia a questo decreto-legge e alla fiducia al Governo, ma anche al termine dell'audizione del Presidente del Consiglio su questa materia, una nota pubblica, in cui sollecita il Parlamento a modificare la normativa introdotta - aggiungo, a titolo personale, con il favore delle tenebre - che modifica e stravolge l'equilibrio tra i poteri e che rappresenta un *vulnus* istituzionale di estrema gravità, che può rappresentare un precedente pericoloso per chiunque poi governerà questo Paese. Mi riferisco e ci riferiamo a quanto, nottetempo e segretamente, è stato introdotto nel decreto-legge,

anche in questa legislatura è stato concesso che, almeno in un ramo del Parlamento, gli emendamenti fossero esaminati. È stata invece introdotta una modifica al titolo,

non è urgente per lo stato d'emergenza, ma nel contempo - udite udite, colleghi parlamentari - della disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica. Questo decreto-legge, cioè, modifica e stravolge gli equilibri tra i poteri dello Stato, modificando i criteri di nomina dei direttori dei servizi segreti, con un atto d'imperio del Governo che infrange il metodo e lo spirito con cui era stata realizzata la legge istitutiva, la n. 124 del 2007. Mi riferisco allo spirito di condivisione a cui si richiama espressamente con un comunicato all'unanimità il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, invitando il Parlamento a ripristinarlo in questa materia, perché, nel campo della normativa sui servizi segreti, è di straordinaria importanza e mi stupisco che i parlamentari entrati in quest'Aula con la bandiera della trasparenza non si rendano conto di cosa stiamo parlando. Che questo sia stato fatto all'insaputa del Parlamento, con una violazione, che credo sia anche costituzionalmente da sanzionare, dello spirito di leale collaborazione tra gli organi istituzionali, Governo e Parlamento, lo testimoniano gli atti avvenuti in Il giorno 28 luglio, in questa sede, il Presidente del Consiglio, illustrando obiettivi e contenuti del decreto-legge in esame, non ci disse nulla sulla sua volontà di modificare la normativa relativa alla nomina dei vertici dei servizi segreti. Le risoluzioni approvate in quest'Aula e alla Camera dei deputati non hanno dato tale indicazione al Governo, che aveva chiesto un'indicazione al Parlamento - il quale gliel'ha data - ma non ha mantenuto gli impegni presi in Parlamento. Nella notte di mercoledì 28 luglio il Governo ha inserito una normativa che nel metodo e nel merito rappresenta un *vulnus* istituzionale.

il Paese lo apprende soltanto dalla *Gazzetta Ufficiale* quando alcuni giornalisti se ne accorgono. Questo è un *vulnus* particolarmente importante, che va assolutamente

davvero impegnata durante il *lockdown* per reperire nel mondo le mascherine e i respiratori di cui avevamo bisogno, viene nominato presidente di Leonardo (siamo a poche settimane prima, in maggio, nel pieno del *lockdown*); in quel caso non c'è stata l'emergenza di prorogare i vertici dei servizi segreti, anzi stato sostituito anticipatamente con un altro direttore. Come mai questo, che non era così urgente - sì da rinnovare anticipatamente il direttore dell'AISE, che è andato a ricoprire l'incarico di presidente di Leonardo - poche settimane dopo, quando invece il *lockdown* ormai è ridotto, diventa urgente e impellente per il direttore dell'AISI? Le nomine spettano al Governo e nessuno vuole assolutamente incidere su questo; è compito e responsabilità suo, anzi del Presidente del Consiglio, nominare e revocare; sono suoi i pieni poteri di indirizzo sui servizi segreti. Proprio per questo, perché sono suoi i pieni poteri - sia di nomina, sia di revoca, sia di indirizzo - per quanto riguarda i servizi segreti, è il Parlamento a legiferare, non colui che ha i poteri, tanto più con l'arbitrio di un decreto-legge imposto con la fiducia. In tutte le democrazie, l'equilibrio dei Poteri ci dice che più ampio è il potere del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica, in questo caso di nomina, di revoca e di indirizzo sui servizi segreti, più ampio dev'essere il controllo del Parlamento e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che infatti ha legiferato sempre in materia in uno spirito di condivisione. Nel metodo, è un *vulnus* istituzionale che costituisce un pericoloso precedente. Nel merito, il provvedimento modifica il provvedimento modifica le modalità di rinnovo e consente una pluralità di rinnovi. Fino a questo momento, secondo la legge istitutiva, i vertici dei Servizi sono nominati con un mandato di un massimo di quattro anni rinnovabile una sola volta; nella storia, cioè nella prassi di questa Repubblica, fino agli anni del Governo Renzi, tutti i Presidenti del Consiglio hanno dato un mandato pieno di quattro anni mai rinnovato, perché sono sufficienti e tutti li hanno ritenuti tali; si era optato per un mandato pieno di quattro anni, mai rinnovato.

o di sei giorni e può rinnovarli ogni sei giorni o ogni sei mesi, in tal modo violando un principio costituzionale tale per cui qualunque mandato nella pubblica amministrazione dev'essere dato con un tempo congruo per essere esercitato in autonomia e responsabilità. Questo tempo congruo non c'è e potrebbe accadere il caso che, essendo rinnovabile innumerevoli volte, può essere rinnovato sei mesi, poi altri sei e ancora altrettanti, trasformando di fatto i direttori dell'Agenzia in attendenti della Presidenza del Consiglio, danneggiando l'equilibrio dei poteri. Stiamo parlando del potere sui servizi segreti, cioè coloro che agiscono con garanzie funzionali per garantire le istituzioni, la democrazia, la libertà, la sovranità e la sicurezza nazionale. In questo campo, ogni parola è importante e ogni norma è decisiva. Il metodo è ancora più importante del merito. In questo caso, ci sono un *vulnus* istituzionale sul metodo, una ferita nel merito, perché in questo modo trasformiamo in precari i direttori dei Servizi, che dipendono soltanto da figure che rispondono al Presidente del Consiglio. È un equilibrio di poteri che la legge aveva ben definito: non può essere stravolto con un decreto-legge, nella notte, all'insaputa del Parlamento e con un doppio voto di fiducia, che non ci consente di deliberare nel merito. Lo dico non come rappresentante di Fratelli d'Italia, membro del Senato e della democrazia italiana: non possiamo concederlo a nessuno, nemmeno a questo Governo.

che consta di soli tre articoli e un allegato. Si tratta essenzialmente, come sappiamo tutti, dell'estensione fino al 15 ottobre dello stato di emergenza deliberato dal Governo il 31 gennaio in seguito all'epidemia da Coronavirus,

del 2020 era molto incentrato sul contrasto e sulle limitazioni; il decreto-legge n. 33 ha proseguito con un graduale allentamento delle misure di contenimento, in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica.

in ragione dell'evoluzione epidemiologica territoriale, il rapporto tra lo Stato e le Regioni. Quindi, ci stiamo muovendo in una cornice normativa di rango primario.

maggiore protagonismo del Parlamento a prendere decisioni con normative di rango primario, e questo sta avvenendo. Ricordo a tutti che il 28 luglio il presidente del Consiglio Conte, venendo in Senato,

Quel giorno abbiamo votato una risoluzione tale per cui bisogna definire con norma primaria le eventuali misure di limitazione delle libertà fondamentali di contrasto all'epidemia, per superare i rilievi di costituzionalità, devono essere non solo limitate nel tempo, ma anche proporzionate all'andamento dell'epidemia. A me pare che in questo quadro ci stiamo muovendo.

iniziative di solidarietà in favore dei familiari dei medici, la facilitazione per l'acquisto dei dispositivi di protezione, nonché misure straordinarie per la produzione di mascherine.

che equiparava al ricovero ospedaliero l'assenza dal lavoro dei lavoratori con disabilità grave, immunodepressi, con patologie oncologiche o che necessitano di terapie salvavita, che sono molto esposti al contagio, o meglio alle alle conseguenze gravissime che potrebbero avere, se contagiati. Questa norma è scaduta il 31 luglio:

Purtroppo non siamo ancora in gestione ordinaria, perché il mondo è in condizioni straordinarie e solo mantenendo alta la guardia e restando in un'emergenza controllata potremo evitare di di nuovo in condizioni di estrema urgenza. Naturalmente non c'è norma che tenga, se non fare appello all'autocontrollo, al senso civico e alla prudenza dei nostri concittadini, ma questo è stato ampiamente dimostrato nel periodo del *lockdown*. Ora c'è il rispetto delle norme semplici a cui tutti siamo ormai abituati: mascherina, lavaggio delle mani e distanziamento; regole semplici per vincere una grande battaglia. Questa è una proroga temporale dell'emergenza, ma qualitativamente - lo sappiamo tutti - è molto diversa da marzo, aprile e maggio, quando la decisione era di essere limitati, chiusi e controllati, perché ha un'intensità più leggera. Sappiamo tutti purtroppo come sono messi i Paesi vicino a noi, come la Francia e la Gran Bretagna, e anche uno Stato come Israele, che sono i tre in cui i contagi sono più numerosi. L'Italia in questa condizione è messa meglio rispetto ad altri, ma abbiamo imparato che un piccolo virus, invisibile all'occhio umano, può mettere in rilievo tutta la fragilità umana e dobbiamo quindi essere molto attenti Di qui al 15 ottobre penso che il Parlamento tutto debba fare un ragionamento su come proseguire nello stato di emergenza e calibrare le norme che ci portano a un'emergenza controllata. Abbiamo fatto l'abitudine a questo, ma fermiamoci un attimo a pensare: stiamo gestendo un'emergenza controllata e cerchiamo di tornare a una normalità. Ci sono state due novità importanti in questo mese: l'apertura delle scuole e il voto di domenica e lunedì, giorni in cui tanti nostri concittadini e concittadine si sono recati alle urne e hanno votato. Questa è stata una grandissima dimostrazione di democrazia e di affezione del popolo del popolo italiano alla partecipazione democratica, nonostante l'epidemia. Quanto alla scuola, penso che tutti insieme dobbiamo ringraziare i direttori scolastici, i presidi e gli insegnanti, che stanno facendo un lavoro immane

se ci sono cose che non funzionano, le correggeremo come parlamentari, insieme al Governo, e soprattutto dobbiamo mettere tantissimo impegno sull'edilizia scolastica e fare in modo che le nostre scuole siano messe a posto. Nel primo giorno di scuola sono andata in un istituto importante di Roma, il liceo Virgilio, e anche lì ci sono problemi di edilizia scolastica e di messa a posto, nonostante lo sforzo immane della preside e della direttrice, che hanno fatto fare lavori d'estate. Credo che dobbiamo aiutare i presidi e tutta

una classe. Quindi dobbiamo essere vicini a tutte le famiglie che stanno affrontando questo delicato momento. Concludo dicendo che l'Italia sta agendo in maniera molto positiva sulla questione del tracciamento. Dobbiamo fare molto di più sulla medicina territoriale. Dobbiamo tenere insieme scuola e territorio, dobbiamo usare le risorse europee e la settimana prossima affronteremo le linee guida sul *recovery fund*. L'umanità è chiamata ad una grande prova.

di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020, adottato dal Governo in relazione alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza ed alla relativa proroga fino al 15 ottobre 2020. Io credo che l'evoluzione dei dati epidemiologici ci racconti che l'incubo pandemia non è alle nostre spalle. Il virus circola con un elevato livello di contagio e, come ci hanno spiegato gli scienziati e gli esperti, potrebbe far configurare il rischio di una seconda ondata. La fine delle misure di *lockdown* ha portato inevitabilmente in questi mesi ad un rialzo del numero dei contagi che sembrano essere per adesso tenuti sotto controllo. Le misure di *testing*, isolamento e tracciamento stanno dimostrando la loro validità e l'Italia risulta, tra i Paesi occidentali, un esempio per ciò che riguarda la prevenzione e la cura del Covid. Lo abbiamo detto quando finì il *lockdown*: con la fase di convivenza con il virus ciò che abbiamo allestito e preparato nei mesi neri di primavera ora deve essere utile esattamente per questo. Ciò che abbiamo imparato in quei mesi deve impegnarci a non abbassare la guardia per non ripiombare in una nuova fase drammatica. Risulta evidente, infatti, che il principio di precauzione e il contenimento cauto e attento del contagio rappresentano in primo luogo la misura giusta e necessaria per garantire la nostra salute ma costituiscono anche, in secondo luogo, il principale strumento che possiede il nostro Paese per far ripartire al meglio e in sicurezza la nostra economia senza esporci a potenziali, probabili ma dolorose battute d'arresto in futuro. Questa è una necessità assoluta per l'Italia. Gli effetti sull'economia li abbiamo visti e non possiamo permetterci di disperdere gli sforzi messi in campo fino ad oggi. Del resto, il quadro europeo e mondiale della pandemia, con intere Nazioni, quando non continenti interi, alle prese ancora con numeri di contagio elevatissimi, rendono evidente l'opportunità di prorogare modalità che consentano una rapida ed efficace risposta, nell'ottica della massima flessibilità, al mutare delle condizioni epidemiologiche, che è appunto la *ratio* che motiva questo provvedimento che rinnova gli strumenti con cui l'Italia ha contrastato con riconosciuta efficacia, in questi mesi, la difficile sfida. C'è un crescente allarme in Europa: paesi come Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna sono alle prese con una impressionante ripresa del coronavirus, tanto da consigliare l'adozione di provvedimenti emergenziali e anche dei mini *lockdown*. Metà Francia è zona rossa. Torna la paura in Gran Bretagna. ci sono stati 241 morti e 11.000 contagi. In Italia constatiamo da settimane il lento e progressivo incremento di positivi asintomatici, una ripresa dei ricoveri e del numero di deceduti. Ci sono dei focolai diffusi nel Paese e l'età media dei contagiati sta aumentando ed ora è di circa quarantuno anni. Questo vuol dire che evidentemente c'è trasmissione intrafamiliare, cioè il virus passa dai più giovani alle persone più anziane. Questo spiega un certo aumento, lento ma graduale, nelle ospedalizzazioni in Lombardia, Lazio, Campania: un *trend* significativo nelle ultime settimane di contagio. Il tema resta dunque quello della prevenzione, dell'innalzare il livello dell'attenzione, di applicare tutte le norme codificate di sicurezza personale e collettiva, secondo le prescrizioni dei protocolli anti-Covid. Per questi motivi è sorta l'esigenza di prorogare, con un atto normativo primario, l'efficacia delle disposizioni dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020. Oggi si impone però anche una riflessione comune e aggiuntiva, e lo dico per il bene del nostro Paese: troppe volte si è sentito gridare contro lo Stato e contro le misure contenitive del virus, che avrebbero strozzato le libertà individuali e di impresa per una semplice smania o addirittura per un piano di controllo da parte dello Stato. Grida e polemiche miseramente naufragate: senza misure preventive e contenitive il virus ancora sussiste, ancora è pericoloso, ancora fa paura e può scatenare una nuova ondata di contagi, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Non possiamo contrapporre il ragionamento economico al tema della gestione della sicurezza sanitaria, anche perché abbiamo visto come in altri Paesi queste scelte abbiano prodotto risultati negativi. In questo senso la riapertura delle scuole in sicurezza e l'avvio delle attività didattiche hanno rappresentato un evento fondamentale per la ripresa ripresa della vita sociale e democratica del Paese. Con le scuole aperte, riparte una delle istituzioni più importanti della Repubblica, il luogo della conoscenza, dell'educazione, della relazione tra generazioni. Consentitemi di dire che non giova a questo obiettivo il fatto che la scuola abbia finito per configurarsi come il bersaglio perfetto nelle settimane scorse, aprendo così il fianco a pesanti e insopportabili strumentalizzazioni. una gestione partecipata a tutti i livelli, da quello ministeriale a quello territoriale scolastico, anche le difficoltà che man mano si presenteranno potranno essere superate. Restano da affrontare le sfide per il futuro, per una strategia complessiva di maggiore valore, a cominciare dal rilanciare un servizio sanitario pubblico equo ed universalistico, che rappresenta una conquista sociale irrinunciabile per i cittadini, con investimenti mirati negli ospedali, per il personale, per la ricerca. Non solo è necessario un sistema universalistico fortemente governato dal pubblico, ma anche un riorientamento sostanziale verso la sanità pubblica e l'assistenza primaria. Abbiamo davanti altri mesi molto impegnativi. Abbiamo qualche preoccupazione, perché il periodo più favorevole al contenimento sta per concludersi. L'arrivo dell'autunno e la ripresa delle attività più socializzanti possono metterci in una condizione più difficile. Queste sono le preoccupazioni, ma non serve cavalcare paure e allarmismi, e nemmeno negare l'esigenza di avere prudenza, di evitare rischi e soprattutto di evitare e scongiurare quello che abbiamo già provato: questo è il compito dello Stato, questo è il compito delle istituzioni tutte. Ritengo pertanto che nel complesso le proroghe disposte dal decreto-legge in conversione correlate, come già ricordato, alla proroga dello stato di emergenza sono necessarie per fare in modo che il Paese sia pronto ad affrontare un eventuale nuovo picco di contagi. Noi voteremo a favore quindi di questo provvedimento, perché abbiamo il dovere di coniugare diritti fondamentali: istruzione, sicurezza, salute. Dobbiamo assicurare la ripresa delle attività economiche e la riconversione ecologica del nostro Paese, tornando ad essere competitivi, rendendo solida quella crescita occupazionale che stiamo intravedendo e utilizzando al meglio le potenzialità del *recovery fund*.

Presidente, colleghi, membri del Governo, il Partito Democratico voterà a favore della conversione del in uno spirito di piena condivisione della filosofia che ha ispirato il provvedimento in esame e in generale l'azione di contrasto alla pandemia, che si è prodotta nel nostro Paese dalla fine di gennaio, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, con la prima delibera del Consiglio dei ministri, fino ad oggi. Ringrazio molto i colleghi che hanno sentito la necessità di stigmatizzare

del pericolo. C'è infatti un filo sottile, ma evidente, che collega il negazionismo al catastrofismo e spesso vediamo che le stesse forze politiche non si fanno mancare nessuno dei due, ma sono, a giorni alterni, vicine o propense a coccolare i negazionisti oppure profeti di sventure (che per fortuna non si realizzano) e i profeti dell'incompetenza, dell'incapacità dei fallimenti del Governo (che mai si sono verificati dal 31 gennaio ad oggi). Penso che un approccio basato sull'equilibrio, sulla ponderazione, sulla flessibilità e sul rigore sia un approccio giusto oggi, come lo è stato in passato e penso che anche il dibattito sull'utilità di prorogare lo stato di emergenza sia stato spesso venato da uno spirito polemico fazioso e da alcune controversie gratuite. Certamente oggi la situazione è meno grave dei mesi di marzo ed aprile, però non possiamo dire che siano scomparsi i pericoli. Ci sono ancora molti rischi dei quali dobbiamo tenere conto e serve ancora una grande prudenza, prudenza, che si riflette nella necessità di dotarci di una apparato decisionale, che possa seguire anche vie non ordinarie, per l'appunto da stato di emergenza. È esclusivamente questa la ragione per cui si propone una proroga e si è fatta una proroga, con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio, "coperta" dal decreto-legge emanato il 30 luglio scorso, quindi il giorno successivo. Non mi sento di condividere nemmeno le critiche che sono state rivolte alla maggioranza e al Governo per il metodo che si è seguito durante questa emergenza. sia stato un metodo corretto e che non ci sia mai stata nessuna volontà di non tener conto e di scavalcare il Parlamento. Abbiamo ad un certo punto ravvisato, nella conversione di un decreto-legge, l'opportunità di mettere nero su bianco la necessità che il Governo venisse con puntualità a rendicontare i risultati della propria azione e i propri intendimenti Da quel momento ciò è puntualmente avvenuto e continuerà ad avvenire, permettendo di arricchire la discussione che si svolge tra di noi, nei vertici delle nostre istituzioni, istituzioni, e di attivare un confronto tra maggioranza e minoranza e tra Governo e Parlamento, che sicuramente ha dato dei risultati importanti, quando lo si è voluto praticare senza faziosità e senza settarismi. Mi pare anche che ci siano state delle prove che siamo riusciti, come Paese, grazie al senso di responsabilità dei cittadini, delle famiglie e delle imprese (ad

efficace, senza traumi e senza sbandamenti e senza che avvenisse nessuno di quei disastri e di quelle situazioni di caos

con la capacità da parte del sistema scolastico nel suo complesso di garantire un buon servizio alle famiglie e ai ragazzi e condizioni di sicurezza certamente idonee. La situazione è destinata a migliorare nelle prossime settimane. Credo che dobbiamo migliorare ciò che ancora non va come vorremmo, ma dobbiamo dobbiamo anche riconoscere che si è lavorato con serietà, in un periodo non facile, durante l'estate, con molte scadenze che pressavano i decisori politici e con i dirigenti delle scuole messi sotto pressione da un susseguirsi di polemiche, di proteste e di preoccupazioni, che non sono proprio il massimo per lavorare in sicurezza. Lo stesso mi pare sia avvenuto per per l'organizzazione delle elezioni: quante ne abbiamo lette di previsioni non nere, ma nerissime? Si è detto che si sarebbe compromesso l'esercizio di un diritto fondamentale, che avremmo compromesso la possibilità dei cittadini di esprimere democraticamente le proprie idee, che non saremmo stati in grado di garantire un flusso ordinato e in sicurezza ai seggi, che sarebbe successo il finimondo. E' successo invece che l'affluenza è stata, in questo turno di elezioni regionali, una delle più alte degli ultimi tempi. Si è votato in due giorni e si è votato in maniera tranquilla e ordinata, come deve avvenire in un grande Paese, con istituzioni perfettamente in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di assolvere ai doveri che sono propri di chi è chiamato a far funzionare la democrazia. Penso che di queste cose si debba tenere conto e penso che si debba continuare a lavorare

dichiarazione di voto a favore su un provvedimento di questa natura, sia il caso di rivolgere un appello forte a tutti coloro che ricoprono incarichi politici affinché non si presti assolutamente nessun tipo di

collegate ad alcuni candidati presidenti, liste che contengono negazionisti del virus, che dicono che in Italia c'è la dittatura sanitaria e che, oltre a questo, servirebbe anche l'Italexit. *(Applausi)*. Bisogna mettersi d'accordo con se stessi. Lo dico senza

perché si mandano segnali sbagliatissimi ai cittadini e si indebolisce il fronte di una lotta complessiva alla pandemia che deve vederci uniti come Paese e determinati a dare il meglio, come Italia e come italiani. Penso che i dati di questi giorni, che dimostrano che siamo in grado, molto più di tutte le altre grandi democrazie europee, di tenere sotto controllo il ritorno di fiamma del contagio, che sapevamo sarebbe stato tra noi dopo l'estate, ci esortino a continuare su questa strada, con serietà e con spirito costruttivo.

Lo siamo perché era nata, subito dopo la fine del cosiddetto *lockdown*, una sorta di promessa - poi rimangiata nei fatti - di collaborazione e comunque sia di attenzione nei confronti delle istanze e delle proposte che l'opposizione portava avanti. avanti. Noi ci siamo quindi attenuti alle parole del Presidente del Consiglio, ma anche delle forze di maggioranza, e alla prova dei fatti, al di là di tutte le questioni di fiducia che sono state messe su provvedimenti che valgono non so bene quante manovre di bilancio, almeno sulla proroga dello stato di emergenza ci saremmo aspettati di poter fare una discussione; contingentata, per carità, con i tempi che si ritenevano necessari, però almeno basata sulla parte relativa agli emendamenti. Per noi è una cosa scontata, ma per i cittadini un po' meno,

così corposi o complessi dal punto di vista economico e finanziario, che si può dare effettivamente un apporto, perché altrimenti non comprendiamo come le forze di maggioranza, il Governo e il Presidente del Consiglio possano ricevere un apporto dall'opposizione. Ci sembra una cosa che dimostra

non si riesce a venire in realtà a capo di nulla. Io mi auguro, anzi lo dico come monito, che questa scenografia non si ripeta sulla questione del *recovery fund*, perché fino ad oggi - ho fatto un controllo stamattina e lo vorrei sottolineare, perché è una questione importante - ho visto apparire semplicemente delle pagine colorate in blu, con delle linee che sarebbero un atto,

quindi con molta franchezza: cerchiamo di capire che il cosiddetto apporto lo si può dare, ma lo si può dare nel momento in cui quantomeno abbiamo delle linee guida abbastanza elastiche non supportate da un orientamento preciso. Quindi, l'attuale questione di fiducia è fiducia è peggiore rispetto alle altre, per il contesto all'interno del quale si è composta, è nata ed è cresciuta, soprattutto perché nasceva

poi così straordinariamente solida questa maggioranza. Io non mi dimentico che nella prima fiducia alla Camera ci fu quel balletto relativo proprio alle cose che ricordava il collega Urso, cioè alla questione della proroga dei vertici dei servizi segreti. Quindi, direi che la situazione non è sicuramente delle più confacenti. Detto questo,

che la faccenda del Covid-19 sia una specie di cosa inventata o esagerata, che serve esclusivamente a "tenere sotto"

quello relativo al modo con cui il sentimento popolare vive lo stato di emergenza, vive le notizie che sono date dai telegiornali e vive la diffusione di quello che viene detto detto con riferimento ai contagi. È un sentimento. Per carità, sta poi in capo alla politica misurare i sentimenti, ma, indipendentemente da questo, sono evidentemente sentimenti che le modalità con cui è stata gestita l'emergenza, e quindi la privazione delle libertà personali, hanno determinato senza che fosse necessaria la spinta o il messaggio di nessuno. nessuno. Attenzione, dunque, alle proroghe dello stato di emergenza che non sono comunque veicolate e spiegate, soprattutto se poi vengono approvate a colpi di fiducia, quindi evitando di fatto

coltivata perché, a suo tempo, crea anche delle ulteriori reazioni di asocialità da parte delle persone comuni e normali.

Siamo di fronte, infatti, ad un Parlamento delegittimato, non solo per l'esito del *referendum*, con cui gli elettori hanno confermato che un terzo di noi non dovrebbe più essere qui, bensì perché il partito che occupa un terzo dei seggi del Senato lo fa in modo abusivo, avendo ormai meno del 10 per cento dei voti del Paese! Ci troviamo, ancora una volta, a votare la conversione di un decreto-legge, dopo che è stato approvato con la fiducia alla Camera e dopo un rapidissimo passaggio in Commissione, senza alcuna possibilità di intervento, anche a fronte di emendamenti di assoluto buonsenso. Questo ramo del Parlamento dovrà digerire questo provvedimento e farlo in fretta, perché siamo a poche ore dalla sua decadenza. Questa è la tanto sbandierata democrazia del MoVimento 5 Stelle anzi, scusate, forse dovrei usare il nuovo nome: Movimento 5 in esame non votiamo, come qualcuno vorrebbe far credere, la proroga dello stato di emergenza; quella l'ha già stabilita il Governo a fine luglio: questo decreto-legge permette invece a Giuseppe Conte di continuare a limitare le libertà costituzionalmente garantite tramite atti amministrativi. Anche se non è quello che viene posto alla nostra attenzione, molto ci sarebbe da dire anche sulla proroga dello stato di emergenza. Nel nostro Paese non c'è più, per fortuna, un'emergenza sanitaria come quando, nella scorsa primavera, gli ospedali erano in *stress* gestionale. L'incremento dei positivi registrato nelle ultime settimane è per lo più dato da soggetti asintomatici che emergono grazie al maggior numero di tamponi effettuati. il minimale aumento di malati e di decessi, che nessuno nega, è tale da giustificare lo stato di emergenza in modo maggiore rispetto ai morti di infarto, di tumore o di incidente stradale? Perché, allora, non dichiariamo lo stato di emergenza anche per queste categorie? L'unica inconfutabile emergenza è data dalla vostra incapacità di gestire la situazione, dalla vostra incapacità di gestire la crisi economica, dalla vostra incapacità di predisporre un piano nazionale per l'autunno, dalla vostra incapacità di gestire la scuola! Non siete capaci nemmeno di fornire le mascherine agli scrutatori ai seggi. *(Applausi)*. Arcuri e Lamorgese le hanno dovute chiedere in prestito alle Regioni per poi, forse, restituirle quando arriveranno quelle che hanno comprato per le elezioni. Vergognatevi!

uno strumento inadeguato, come sottolineato più volte da tantissimi costituzionalisti. Come abbiamo ripetuto più volte, si tratta di un mero atto amministrativo di rango secondario che non potrebbe assolutamente interferire sulle libertà di movimento, di riunione, di religione e di impresa, come invece avvenuto negli ultimi mesi. La nostra Costituzione prevede, all'articolo 77, uno specifico strumento legislativo da adottare in condizioni di necessità e di urgenza: il decreto legge, che è sottoposto al vaglio del Capo dello Stato (proprio per la sua importanza di intervento in situazioni straordinarie) e, soprattutto, a quello del Parlamento (deputato alla sua conversione). La nostra Costituzione prevede quindi, anche in casi straordinari e urgenti, un ruolo attivo del Parlamento per garantire l'equilibrio tra i poteri. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplici atti normativi secondari e, come tali, non solo sono sottratti al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica, ma sono insindacabili anche *ex post*, in quanto sfuggono al controllo successivo della Corte costituzionale. hanno invece inciso in maniera rilevante sui diritti inviolabili e sulle libertà fondamentali di ogni individuo e della collettività, fino a giungere a comprimerli completamente e continueranno a farlo per tutto il tempo della proroga che si vuole concedere il provvedimento contravviene anche all'impegno che il Governo aveva assunto solennemente dinanzi al Parlamento, in virtù del quale si era impegnato ad adottare eventuali nuove misure limitative o sospensive delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili previsti e tutelati dalla Costituzione con legge o atto avente forza di legge. Solo con quelli! *(Applausi)*. Il decreto-legge in esame, prorogando le norme emergenziali, contribuisce oltretutto ad aumentare un clima di tensione che incide negativamente sull'economia nazionale. Bisognerebbe concentrare l'attenzione su poche e semplici norme di prevenzione (mascherine, distanziamento e igiene), sul ritorno graduale e prudente alla normalità e sul rilancio dell'economia e delle imprese.

Ma se, come dite, lo stato di emergenza è davvero così necessario, perché continuate a permettere e ad incentivare gli ingressi illegali nel nostro Paese? Ma certo, garantite per tutti i clandestini tutti i controlli, tamponi rapidissimi, assistenza sanitaria, luoghi confortevoli e navi di lusso dove trascorrere la quarantena, tutte cose che però non siete in grado di garantire agli italiani. Prima lo straniero, prima il clandestino, questo è il vostro motto! *(Applausi)*. Avete fatto quadruplicare gli sbarchi, con lo scopo di assicurare quella che per voi è la vera emergenza politica: quella di far riprendere il *business* dello sfruttamento, il *business* dell'accoglienza, il *business* del caporalato e della schiavitù, il *business* della malavita, senza contare senza contare i tantissimi ingressi che non siete in grado di controllare, come ad esempio quelli della pista balcanica. Così facendo, state mettendo a rischio la salute dei cittadini, siete degli irresponsabili e prima o poi ne dovrete rendere conto. Siete così attenti a pensare ai clandestini che vi siete dimenticati di una fetta di connazionali tanto importante quanto estremamente delicata, quella dei lavoratori fragili, degli immunodepressi e di coloro che sono tutelati dalla legge n. Fino a fine luglio, i decreti precedenti avevano previsto una tutela per queste categorie fortemente a rischio, che lo sono tutt'ora, anche di fronte ad una carica virale limitata come quella in circolazione in momento. Ve ne siete dimenticati. Avete detto a queste persone: «Andate in fabbrica, andate sul treno, andate sul tram; anzi, attaccatevi al tram: per voi i soldi non li abbiamo stanziati, perché stiamo ancora facendo i calcoli dell'impegno di spesa, però se volete vi regaliamo un monopattino». *(Applausi)*. Questo gli avete detto. Li state esponendo ad un rischio inutile, ve ne rendete conto? Concludo, Presidente, toccando un tema estremamente delicato, il comma 6 dell'articolo 1, che va a modificare le modalità di rinnovo dei vertici dei servizi segreti, una disposizione estremamente grave per tre motivi. Il primo è che non vi è stata alcuna anticipazione del dibattito parlamentare e non c'è stato alcun confronto con le forze d'opposizione, cosa che dovrebbe essere sacrosanta quando si interviene sui cardini delle garanzie repubblicane e su una legge che, come in questo caso, era stata approvata con la condivisione di tutto l'arco costituzionale. Il secondo è che si va a limitare l'autonomia dei vertici dei Servizi dando a Conte un potere che nessun altro Presidente del Consiglio ha avuto negli ultimi ottant'anni. Lo stesso Copasir ha richiesto una modifica perché si intervenga quantomeno per definire per definire tempi e modalità delle proroghe. Questo fatto gli è stato ricordato anche questa mattina dal senatore Arrigoni, ma voi fate orecchie da mercante e tirate dritto su un testo che - lo sappiamo tutti - è inviso anche a gran parte della vostra maggioranza. terzo è che non vi è alcuna ragione di inserirla in un provvedimento come questo, che tratta tutt'altro e che per il principio di omogeneità del decreto avrebbe dovuto essere stralciata. È una vera e propria forzatura, che pone degli interrogativi molto pesanti. Se c'è un nesso tra servizi segreti e Covid, adesso ci dite qual è. *(Applausi)*. La casa della democrazia, questo Parlamento, deve essere di vetro, deve essere trasparente, non può esserci nemmeno il minimo dubbio che qualcosa di poco chiaro sia accaduto, magari nei rapporti con una potenza straniera orientale. E questo non è l'unico punto oscuro: ci sono i verbali del comitato tecnico-scientifico sulle zone rosse, resi pubblici in ritardo e solo parzialmente e ci sono i *dossier* sulle previsioni della pandemia tenuti segreti e di cui non venne data informazione alle autorità sanitarie e ai governatori delle Regioni. Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova, la prova che gli italiani stanno pagando un conto troppo caro ad un *Premier* e al suo movimento che ad ogni elezione viene umiliato dal voto popolare. Per tutti questi motivi, Presidente, il Gruppo Lega Salvini Premier non voterà la fiducia a questo Governo.

Signor Presidente, colleghi, all'indomani della prima ondata di emergenza il 74 per cento degli italiani giudicava positivamente il modo con cui il Governo aveva gestito la crisi da coronavirus; uno dei valori più alti fra le grandi economie avanzate, secondo quanto riportato da un sondaggio condotto in 14 Paesi dal Pew Research Center.

la Spagna registrava quasi 10.000 casi al giorno e l'Italia più di 6.500; entrambi i Paesi hanno riportato la situazione sotto controllo con una combinazione di *leadership,* umiltà, partecipazione attiva di ogni membro della società e un approccio globale; entrambi i Paesi hanno affrontato una situazione scoraggiante, ma l'hanno capovolta; lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità in conferenza stampa a Ginevra. Di questa corretta gestione stiamo sentendo ancora oggi le ricadute positive: mentre gli altri Paesi sono quasi vicini a nuove chiusure, in Italia si sono tranquillamente potute tenere le consultazioni elettorali e l'indice RT è ancora oggi fra i più bassi d'Europa. L'emergenza non è conclusa e anzi ci prepariamo ad un periodo non facile in cui sarà importantissimo agire beneficiando di quanto abbiamo appreso nei mesi trascorsi. Abbiamo tutti il dovere di non vanificare gli effetti positivi ottenuti grazie ai sacrifici enormi che i cittadini italiani hanno compiuto, con un senso di responsabilità che ha in parte stupito il mondo ma che ci viene oggi riconosciuto. Contenere Contenere e contrastare l'emergenza rimangono azioni imperative per preservare la salute dei cittadini, pure alla luce del graduale e giusto allentamento delle misure più restrittive che abbiamo conosciuto nei mesi scorsi. La pandemia è un processo in continua evoluzione, tale da richiedere la massima prudenza possibile. La situazione del resto del mondo è ancora drammatica e presenta anche in Europa un quadro epidemiologico particolarmente deteriorato. La centralità del Parlamento nel definire le linee di indirizzo nella gestione della fase emergenziale è indiscussa. Nel rapporto tra Governo e Camere occorre ricordare che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato devono illustrare preventivamente il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tener conto, così come è stato fatto, di eventuali indirizzi dalle stesse formulati e, ove non sia possibile per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure adottate, comunque il Governo riferisce successivamente. Superata quindi l'*impasse* creatasi nel primo periodo, dovuta non certo alla malafede ma alla concitazione e alla gravità del momento, mi appello a tutti affinché si possa agire con la massima fiducia e collaborazione. Ho sentito polemiche sterili anche in relazione ai rapporti tra Presidente del Consiglio e servizi segreti (le abbiamo ascoltate poc'anzi); l'audizione di ieri, durata oltre due ore, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte presso il Copasir va nella medesima direzione di trasparenza istituzionale a cui il Governo si è sempre attenuto; qualora dovessero emergere criticità, così come affermato dallo stesso Copasir in un comunicato a margine dell'audizione, l'obiettivo sarà quello di intervenire sulle norme della legge n. 124 del 2007 in materia di nomina dei direttori delle agenzie di informazione e sicurezza, in uno spirito di collaborazione che non può e non deve mancare. Oltre a questo, è comunque emersa l'esigenza, superando le logiche emergenziali e contingenti, di avviare quanto prima un'organica azione di aggiornamento della legge stessa, al fine di adeguarla all'evoluzione del quadro istituzionale e alle nuove minacce per la sicurezza. basta con illazioni infondate, che non fanno bene al nostro Paese, che ora ha ben altre priorità. È sotto gli occhi di tutti la trasparenza con cui questo Governo sta agendo e continuerà a farlo, così come è ben chiara la vostra costante volontà di delegittimare il lavoro svolto dal presidente Conte e da questa maggioranza. Il nostro Governo ha sempre agito nell'esclusivo interesse della salute di tutti noi. Oggi siamo chiamati a garantire continuità alla condotta dell'Esecutivo che, guidato da principi di adeguatezza e proporzionalità, ha permesso di adottare azioni fondamentali di assistenza ai cittadini, così come interverrà nella tutela dei lavoratori fragili, che rappresenta una priorità di questo Parlamento e di tutto il Governo. Il provvedimento che stiamo votando, dunque, è questo, abbiamo tutti il dovere di ribadirlo: non significa andare verso un nuovo *lockdown*, ma esattamente il contrario. Stiamo lavorando per impedire in maniera preventiva che ciò possa avvenire. Mi avvio alla conclusione, Presidente. I numeri in Italia e nel mondo e l'assenza di un vaccino o di un'efficace terapia farmacologica ci dicono che non possiamo abbandonare il senso di responsabilità che ci ha guidati finora. La proroga dello stato di emergenza è una scelta dettata dal bisogno di sicurezza che si impone in un Paese che si vuole avviare gradualmente alla normalità; è un passaggio determinante che incide su questioni cruciali per la comunità. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indìco pertanto tale votazione. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto,

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1928, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,

Signor Presidente, intervengo relativamente all'interrogazione

nel quale i rappresentanti di 150 Comuni lamentavano il fatto che in moltissime aree, soprattutto nelle zone montane, pedemontane e collinari, il segnale Rai arrivava praticamente mai o in modo molto sporadico. A seguito di quella segnalazione, tra l'altro riguardante circa 300.000 abitanti in Piemonte, la Rai interveniva comunicando che dai dati in suo possesso

che vorremmo vedere nei fatti adempiuto quell'impegno preso all'inizio del 2019, e cioè il 100 per cento di copertura del segnale Rai, che tra le altre cose è un diritto esplicito dei cittadini che giustamente lo stanno rivendicando.

nei giorni scorsi ho rivolto pubblicamente un appello al ministro Franceschini, nella convinzione che la sua distrazione rispetto a un gravissimo fenomeno in corso non sia ulteriormente tollerabile. Mi riferisco alle demolizioni che soprattutto in Campania, complice il cosiddetto piano casa, ma anche altrove sull'intero territorio nazionale, stanno interessando l'edilizia storica di età rinascimentale e moderna fino al XIX secolo, sia nei centri urbani sia nelle campagne. fuori e dentro le nostre città complessi monumentali di eccellente qualità architettonica, non di rado pluristratificati, finiscono letteralmente in polvere, anche in una sola giornata di lavoro data la potenza degli escavatori disponibili, per far posto a lottizzazioni che potrebbero tranquillamente sorgere altrove senza questo immane sacrificio. Troppo spesso l'abbandono di edifici e complessi edilizi storici è sufficiente, insieme alla ruderizzazione più o meno avanzata, per giustificare l'abbattimento sconsiderato di questi pezzi

chiamati a intervenire in emergenza, demolendo, su strutture di cui ignorano le reali condizioni di stabilità. Spetta al Parlamento avviare finalmente la discussione della proposta di legge sui centri storici che si deve all'associazione Bianchi Bandinelli, e in questi giorni sembra finalmente muoversi qualcosa in questo senso. Ma un Ministro della cultura - per parte sua - non dovrebbe assistere a uno spettacolo così drammatico senza tentare con ogni mezzo a sua disposizione di porvi un freno e soprattutto tacendo. tacendo. Proprio oggi, leggevo su «La Prealpina» che, dopo aver ragionato sul punto con il ministro Bellanova, Franceschini auspica un intervento tipo ecobonus per i casali di campagna perché - cito alla lettera - «è un dolore vedere casali meravigliosi abbandonati o crollati». Una prospettiva meramente estetizzante, sentimentalistica, che credevamo superata da decenni, è il solo sentimento che il titolare del Mibact riesca a manifestare, e sia pure, purché serva a salvare quel patrimonio edilizio senza stravolgerlo, e sottolineo senza stravolgerlo. Più concretamente, però, Presidente, mi permetto di affermare che è necessario - e non può attendere oltre - un censimento dell'edilizia storica su tutto il territorio nazionale, sia urbana sia rurale, che al più presto fornisca agli uffici territoriali del Mibact i dati utili a valutare l'opportunità di avviare verifiche dell'interesse culturale e conseguenti vincoli. Ne va della nostra memoria nazionale materializzata nel paesaggio italiano, tanto decantato anche all'estero. Prima di digitalizzare il patrimonio, con tutto il rispetto per una simile iniziativa, anch'essa sponsorizzata nei giorni scorsi, quel patrimonio va difeso, altrimenti molto presto non ci sarà più alcunché da digitalizzare né alcuna identità nazionale in cui riconoscersi.

il Conte-*bis*, non si vedono ancora iniziative, si sentono solo mere dichiarazioni di intenti. Ricordiamo che il regionalismo differenziato è una grande opportunità, una soluzione per un riassetto generale di uno Stato la cui debolezza istituzionale è ormai nota da tempo e che si è palesata veramente in modo drammatico durante questa emergenza sanitaria. Il regionalismo differenziato è sostanzialmente la valorizzazione di eccellenze e di caratteristiche locali, è responsabilità della politica locale: hai delle competenze, le devi gestire bene. Noi avevamo proposto un impianto; abbiamo fatto più di un centinaio di incontri per la trattativa con le Regioni e con i vari Ministeri: usate quel lavoro senza perdere ulteriore tempo. Il meccanismo di finanziamento, che avevamo elaborato con il superamento della spesa storica verso i fabbisogni *standard,* consente, sì, di gestire le risorse, ma impone altresì alle Regioni quell'efficientamento che oggi è indispensabile per far sì che questa nostra Italia sia finalmente competitiva e abbia il futuro che merita un grande Paese come il nostro. Ricordate che il regionalismo non nasce nelle segrete stanze di qualche sede di partito - e questo lo dico anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - ma nasce nel e fra il il popolo. Abbiamo appena adesso celebrato un *referendum*, l'ultimo. I risultati dei *referendum* non si commentano: semplicemente si rispettano e si eseguono. Abbiamo indetto un *referendum* in Veneto e in Lombardia:

E se in Veneto il presidente Zaia ha avuto un consenso che si è attestato al 76,79 per cento, con un programma che vede l'autonomia e la richiesta di autonomia al primo posto,

Signor Presidente, come Gruppo Forza Italia abbiamo da poco depositato un'interrogazione parlamentare perché è evidente che il diritto di viaggiare con adeguati *standard* di servizio, uguali su tutto il territorio nazionale, è un lusso del quale i cittadini calabresi non possono godere. Il Governo è responsabile quanto Trenitalia della sempre maggiore distanza tra la Calabria e il resto d'Italia e le oltre sei ore di viaggio che, dal 21 settembre scorso fino - si spera al 12 ottobre, gli utenti dovranno sopportare per percorrere il tragitto Reggio Calabria-Roma e Roma-Reggio Calabria ne è solo un esempio lampante. Una presenza di collegamenti efficiente è il punto di partenza imprescindibile per lo sviluppo turistico e commerciale di un territorio. Il ricordo del *premier* Conte che lo scorso 14 febbraio annunciava a Gioia Tauro la diminuzione a quattro ore del tempo di percorrenza dei treni tra Roma e Reggio e Reggio e Roma è ancora nitido nella mia mente, così come sono ben chiare nella mia mente le pagine del Piano Sud 2030, sviluppo e coesione per l'Italia. Tenga questo Governo fede ai propri impegni con la Calabria e faccia partire quanto prima i cantieri per portare la vera Alta Velocità anche a Sud di Salerno. Non possono continuare ad esistere due Italie: una collegata con infrastrutture moderne ed efficienti e un'altra in cui bastano dei semplici lavori per tornare agli anni Sessanta. Presidente, colleghi senatori, è chiaro però, purtroppo, come il vagone su cui viaggia questo Esecutivo sia in ingiustificabile ritardo. Per questo chiedo al Governo e ai Ministri interrogati di rispondere nel più breve tempo possibile, dando certezza della conclusione dei lavori entro la data annunciata e intraprendendo azioni concrete al fine di tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini calabresi, nonché dei turisti che vorrebbero visitare i nostri splendidi luoghi viaggiando su treni mediamente veloci, puliti e a costi non eccessivamente alti.

apre una nuova finestra"). Vorrei richiamare l'attenzione su una questione inerente lo stato di disagio in cui versano centinaia di lavoratori delle ex agenzie di recapito che oggi sono privi di occupazione, nonostante per decenni queste ultime abbiano svolto attività di recapito di tutti i prodotti postali sull'intero territorio in regime concessorio. Ripercorrendo brevemente la normativa di riferimento, si osserva che con il decreto legislativo n. 261 del 1999, di recepimento della direttiva 97/67 della Comunità europea, erano state revocate le concessioni alle agenzie di recapito, prevedendo l'introduzione degli istituti della licenza individuale e dell'autorizzazione generale per lo svolgimento dei servizi postali non riservati. Si è registrata dunque una progressiva e inesorabile riduzione dei livelli di occupazione all'interno delle agenzie di recapito, le quali hanno visto ridurre il loro numero da 70 nel 2000 a 10 nell'ultimo periodo. Con un primo atto di sindacato ispettivo del'11 ottobre 2018 avevo già evidenziato la problematica *de quo*. Successivamente alle mie iniziative era stato aperto presso il Mise un tavolo di confronto con Poste italiane per la ricollocazione degli ex lavoratori. tenutosi al Mise, Poste italiane aveva manifestato l'intenzione di procedere alla suddetta ricollocazione previa consegna di un elenco con i nominativi dei lavoratori interessati e iscrizione nella sezione «lavora con noi» sul sito della stessa società. Nonostante l'inoltro Nonostante l'inoltro del predetto elenco, in data 19 luglio 2019 non risulta essere stata attivata alcuna procedura di chiamata e, quindi, sulla problematica ho predisposto un altro atto di sindacato ispettivo di cui ho dato sollecito. Spero veramente che il Governo prenda in carico questa problematica e che Poste italiane possa risolvere la questione.